la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 marzo. Nella seduta di oggi si svolgerà la discussione generale sul decreto-legge proroga termini. Le repliche e le votazioni si terranno nella seduta di domani. L'ordine del giorno della seduta di domani prevede, inoltre, la discussione, dalla sede redigente, del disegno di legge recante introduzione del reato di omicidio nautico e delle ratifiche di accordi internazionali per le quali l'Assemblea ha accolto la procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Giovedì mattina, alle ore 10, avrà luogo la chiama per la votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di tre senatori Segretari. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 12. Seguiranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time* con la presenza dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali. Il calendario della prossima settimana prevede l'esame dei seguenti argomenti: decreto-legge in materia di impianti di interesse strategico nazionale; deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento per il disegno di legge recante modifiche alle disposizioni per il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali; decreto-legge sulla gestione dei flussi migratori, attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati. Il calendario della settimana sarà integrato con le votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria. tributaria. Nella settimana dal 28 febbraio al 2 marzo si discuteranno il decreto-legge sulla ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e, qualora nel frattempo sia deliberata la procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, il disegno di legge sulle modifiche alle disposizioni per il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali. Il calendario della settimana dal 7 al 9 marzo prevede la discussione del decreto-legge sulla trasparenza del prezzo dei carburanti, in corso di esame presso la Camera dei deputati, e, ove concluso dalla Commissione, del disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

che sicuramente in cuor loro hanno qualcuna o qualcuno a cui esternano tutta la loro amicizia e il loro amore. Buon san Valentino a tutti. *(Applausi)*.

credo di dover esprimere innanzitutto un ringraziamento vero, sostanziale e non formale a tutta la Commissione, a tutti i componenti della 1a e della 5a Commissione perché siamo riusciti siamo riusciti a esaminare un provvedimento complesso come quello odierno entrando nel merito, vagliando più di trecento emendamenti, cinquanta audizioni in presenza, con oltre quaranta contributi scritti. Credo sia stata la prima volta che sul mille proroghe si siano fatte audizioni. È stato un lavoro utile e fruttuoso. Sono venuti tantissimi spunti, che poi i Gruppi hanno trasformato in emendamenti. Il Governo, anche su sollecitazione mia e del collega senatore Calandrini, ha preso l'impegno, che ha poi mantenuto, di non presentare emendamenti sulle stesse materie sulle quali insistevano già emendamenti di iniziativa parlamentare, non importa se di maggioranza o di opposizione. Credo Credo quindi che abbiamo fatto un lavoro molto importante. Certamente non siamo riusciti ad accogliere tutte le proposte che pure avrebbero meritato di essere approvate. se andate a esaminare i lavori delle nostre due Commissioni, scoprirete che sono stati approvati tantissimi emendamenti di iniziativa parlamentare, sia di maggioranza che di opposizione. C'è stato quindi un confronto molto costruttivo, che ci consegna un testo A certamente più ricco

sono stati gli emendamenti presentati per l'Assemblea. L'impegno era di contenerne il numero a poche questioni essenziali: vedo che il numero non è proprio così contenuto, perché siamo ad oltre 200 emendamenti. Tuttavia, con un po' di buona volontà, se lavoriamo bene, anche in Assemblea credo che saremo in grado, grazie anche al lavoro del Governo, di concludere i nostri lavori così come li abbiamo iniziati, cioè in un clima costruttivo e di collaborazione. Ringrazio tutti e auguro buon lavoro.

vedeva anche le aspettative dei Gruppi parlamentari. Abbiamo fatto il massimo senza alcune risorse e senza *plafond* e ci eravamo dati un percorso: volevamo oggi, con questo decreto-legge, cercare di rispettare

alcuni interventi sull'università, sugli ordini professionali e soprattutto sulla questione delle costruzioni, prevedendo la possibilità di accordi quadro e di prezziari per quanto riguarda il caro materiale, che in questo momento sta mettendo in seria difficoltà i cantieri e i lavori pubblici nel nostro Paese.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà. Signor Presidente, mi ha sempre fatto sorridere il nome di questo decreto-legge: milleproroghe.

nessuno innocente da questo punto di vista. Ma dal punto di vista del diritto - sarà che sono avvocato - mi ha sempre fatto sorridere che questo Paese assuma un tale provvedimento, soprattutto se poi nel provvedimento ci sono delle norme un po' particolari. Io ringrazio - e non lo faccio in modo formale - i presidenti delle Commissioni, Calandrini e Balboni, e il relatore Damiani, per essere stati attenti ascoltatori delle opposizioni. Hanno fatto passare numerosi emendamenti e quindi li ringraziamo. ci lasciano perplessi alcuni emendamenti che sono stati approvati dalla maggioranza. Facciamo un passo indietro. Innanzitutto siamo felici degli emendamenti di Italia Viva approvati (a prima firma mia, della collega Gelmini e del collega Lombardo),

una soluzione alle problematiche aperte. Cito l'emendamento a firma della mia collega Paita, che prevede che le concessionarie autostradali siano obbligate a venire nelle Commissioni parlamentari a esplicitare gli interventi sulla sicurezza nella manutenzione delle autostrade; un emendamento sentito, soprattutto dopo la tragedia del ponte Morandi e non solo.

Mi lasciano più perplessa invece altri emendamenti: il collega relatore ha indicato quello sui balneari. Come possiamo non fotografare cosa è successo in Commissione su quell'emendamento? Una maggioranza molto unita nell'intento di prorogare le concessioni, ma divisa sul modo di scrivere il testo. Ciò è tanto vero che - sarà anche per dar merito a ciascuna delle forze politiche che sostengono il Governo - ci sono ben tre emendamenti sul tema, quando di solito

Decidendo *sine die* di non individuare una soluzione e prorogando tal quale, senza introdurre elementi di novità all'interno dell'emendamento, temiamo di andare incontro a una sanzione europea, con una procedura di infrazione nei confronti del nostro Stato; un'infrazione che pagherebbero tutti i cittadini proprio perché non si è voluto decidere, e mi sembra cosa non corretta e non giusta.

interlocuzione e soprattutto che i tempi di proroga oltre i tre anni fossero un elemento di mancanza di concorrenza. Ci è voluto, appunto, il Quirinale per fare giustizia di un emendamento che tutte le opposizioni - in maniera univoca - avevano considerato fuori luogo, fuori tempo e soprattutto portatore di interessi troppo particolari e soggettivi per essere considerato di interesse nazionale.

rivedere le vostre posizioni non tanto e non solo in merito alle promesse elettorali fatte, che sono legittime, quanto in relazione a soluzioni che possano creare nocumento alla nostra Nazione. Da

al Governo che le hanno suscitato alcune critiche. Da quel momento siamo stati considerati perennemente la quarta gamba del Governo, ma non avete bisogno di avere quattro gambe né noi siamo interessati a essere una gamba. Siamo interessati a fare il bene del Paese e a dire sempre le cose che pensiamo con la schiettezza e la rigorosità che ci appartengono. Aver approvato determinate norme in questo milleproroghe non farà bene al Paese;

non ho molto tempo a disposizione, per cui ho deciso di dedicarlo a un unico punto specifico del decreto-legge in esame. Voglio parlare del FIR, il Fondo indennizzo risparmiatori, il Fondo indennizzo risparmiatori, introdotto con la legge di bilancio del 2019 per compensare i risparmiatori truffati dalle banche. Esso prevedeva l'erogazione di un rimborso del 30 per cento del prezzo di acquisto delle azioni e del 95 per cento del valore delle obbligazioni. Credo si possa affermare che il Fondo, dopo alcuni iniziali problemi di assestamento, ha funzionato bene e ha offerto un minimo di ristoro ai risparmiatori che, in taluni casi, avevano perduto tutto il loro patrimonio. da Consap, il Fondo aveva una dotazione iniziale di 1.575 milioni, che, però - ed è questo in particolare il tema del mio intervento - è stata utilizzata solo in parte. Dai dati finora messi a disposizione pubblicati dal MEF risulta che, al 31 dicembre 2022, il saldo tuttora inutilizzato ammonta a circa 500 milioni di euro. I lavori della commissione tecnica nel frattempo sono stati completati al 31 dicembre scorso e sono stati prorogati, proprio con questo provvedimento che stiamo esaminando, fino al 30 giugno 2023 con il testo originario del decreto-legge e, con un ulteriore emendamento, al 31 dicembre di quest'anno. Abbiamo salutato con favore l'iniziativa del Governo che ha offerto una possibilità di riesame di diverse posizioni oggetto di contenzioso.

ne era peraltro consapevole lo stesso legislatore del 2018, tant'è che fin dall'originaria stesura, al comma 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, era previsto che la percentuale del 30 per cento poteva essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto fossero inferiori alla previsione di spesa. È esattamente quanto è accaduto in quegli anni, tant'è che - come abbiamo detto in premessa - oggi risulta maturato un saldo positivo di 500 milioni. Che cosa vogliamo fare di questi quattrini? È giunto il tempo di prendere una decisione e incrementare proporzionalmente la percentuale degli indennizzi, in conformità alla lettera e allo spirito della legge istitutiva; anche perché i *leader* di tutti i nostri partiti nella campagna elettorale dello scorso autunno hanno preso, pubblicamente e anche per iscritto, degli impegni nei confronti delle associazioni dei risparmiatori. In campagna elettorale le associazioni dei risparmiatori hanno chiesto un impegno e *leader* di pressoché tutti i partiti presenti in quest'Aula hanno risposto di sì e detto che si farà così. A tale proposito, illustre Sottosegretario, la voglio informare che ho predisposto e depositato un ordine del giorno in linea con quanto ho proposto. Nei mesi scorsi alcuni parlamentari sensibili al tema - parlamentari di tutti gli schieramenti, va riconosciuto - avevano tentato di presentare degli emendamenti finalizzati all'incremento dell'indennizzo. Questi emendamenti sono stati tutti o respinti o ritirati su richiesta del Governo. Nelle interlocuzioni informali, la scusa generalmente addotta era il parere contrario del direttore generale del MEF, dottor Rivera. Ho l'impressione che quello fosse solo un alibi. se alibi era, oggi è venuto meno, perché il dottor Rivera non c'è più ed è stato destituito dal suo incarico. Mi aspetto quindi, signor Sottosegretario, un parere favorevole secco sull'ordine del giorno. Capisco che, considerate le ristrettezze di bilancio, al MEF ci possa essere la tentazione di destinare ad altre finalità i fondi del FIR: il Paese è in difficoltà e c'è bisogno di risorse per colmare molti buchi. Ma sarebbe un grave errore. Sarebbe innanzitutto un tradimento degli impegni assunti in campagna elettorale da tutti i *leader* dei partiti presenti in quest'Aula e della fiducia che gli elettori hanno riposto nei loro rappresentanti in Parlamento; soprattutto, costituirebbe un autentico scippo contabile. Mi spiego meglio: i fondi FIR non provengono dalla fiscalità generale, non sono il frutto delle tasse o di *deficit* pubblico, ma sono somme recepite nei conti dormienti delle banche, sono state destinate e messe a disposizione proprio dal sistema bancario per sanare le profonde ferite inferte alla sua credibilità dopo la crisi del 2011. Sottrarle alla loro destinazione originaria e destinarle a fini di fiscalità generale costituirebbe quindi una operazione di dubbia legittimità contabile e costituirebbe anche un pericoloso precedente. Confido che il Governo, ascoltate le mie parole e le mie sollecitazioni, manterrà fede ai suoi impegni ed esprimerà parere favorevole all'incremento della percentuale dell'indennizzo del FIR, come peraltro tutti i nostri *leader* politici hanno promesso in campagna elettorale. *(Applausi)*.

proroghe che sono necessarie fino a un certo punto se fatte in un certo modo. Per i cittadini italiani è infatti necessario e urgente un piano di sviluppo che sia definito e pianificato in un processo costante affinché tutti abbiano il tempo di orientare le attività con aspettative certe. Non può essere l'attesa di una proroga a dare la spinta alla ripresa di tante attività che sono in drammatico affanno e devono urgentemente fare i conti con il proprio futuro. Per strutturarsi in modo utile è necessaria una pianificazione a lungo termine: lo diciamo spesso. Siamo in una fase storica in cui tanti hanno perso tutto e queste proroghe, a parte quelle legate a meri atti d'ufficio, devono servire a dare un segnale di rotta programmatica alle tante attività lavorative in campo; rotta che si fa fatica a leggere e che, purtroppo, spesso è solo un enorme vuoto, un nulla che ci lascia sgomenti. Penso a quanto non fatto per tutto il sistema del *bonus* 110, ai crediti rimasti bloccati nei cassetti fiscali, al settore edile in ginocchio dopo che, invece, finalmente aveva trovato un fulgido sviluppo. È stato come lanciare una bomba su una superstrada. Ora è il caos. Si stanno quantificando i danni. Si sta verificando se si è vivi o morti. per tante attività produttive, per tante realtà lavorative in attesa di percepire un'attenzione del Governo al loro futuro. loro futuro. È necessario dare una direzione certa oggi, ma che guardi al domani. È un punto importantissimo in questo momento in cui tante attività vedono il buio innanzi a sé o una strada molto in salita. Ora voglio focalizzarmi su aspetti relativi alla mia Commissione, la 9ª Commissione, quindi al settore agricolo e della pesca in *primis*. Siamo riusciti a intervenire e inserire un emendamento portato a gran voce un po' da tutti, che è quello per la proroga dei termini di utilizzo dell'incentivo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio agricolo effettuato nel terzo e quarto trimestre del 2022. Conosciamo tutti le fortissime difficoltà legate al caro benzina. di chi vive questo problema, legato a tanti altri che certamente annullano tutto il guadagno, diventa un mero dovere del Governo garantire la possibilità di beneficiare di tale incentivo. Quindi, un credito di imposta per l'acquisto dei carburanti è indispensabile. Oggi portiamo la proroga fino al 30 giugno: una misura ancora più doverosa in quanto non comporta spese aggiuntive. Riguardo la necessità di potenziare i settori promettenti, siamo riusciti a dare un aiuto ai birrifici artigianali, un comparto che si è rivelato particolarmente trainante negli ultimi anni, ma che ha subito una forte battuta di arresto nel periodo pandemico. Tanti, che con entusiasmo hanno intrapreso questa attività produttiva, si sono dunque trovati in seria difficoltà e in questi mesi sono stati con il fiato sospeso, vedendo in scadenza la possibilità di usufruire del taglio delle accise accordato nel precedente Governo. Grazie a un emendamento a mia prima firma per il MoVimento 5 Stelle, abbiamo raggiunto questo obiettivo. Unitamente agli sconti progressivi per i birrifici artigianali, si mettono a disposizione 8,15 milioni di euro per il 2023. La direzione è rendere il sistema italiano attrattivo, dando forza anche ai piccoli produttori, nonché ridare slancio alla filiera, che è sì industriale, ma anche agricola, e così garantire la tenuta occupazionale, essenziale al giorno d'oggi. Utile è la proroga per il triennio 2023-2025 agli incentivi per gli investimenti in colture arboree pluriennali, come olivi, vigneti e frutteti. Trattandosi di di colture caratterizzate da rese che richiedono almeno tre anni di tempo, esse hanno necessità di siffatti incentivi. Ma questo - lo ripeto - deve essere un inizio che deve essere poi perseguito; deve essere un inizio che deve dar vita a delle aspettative per un futuro pianificato in tal senso. È questo che io oggi voglio chiedere al Parlamento e al Governo. Utile è la proroga per la validità dei patentini per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari fino al 30 giugno, per garantire al sistema il tempo necessario a smaltire il grande numero di autorizzazioni in attesa di rinnovo. Abbiamo poi la proroga al 31 dicembre per le misure di intervento straordinario a favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi

posizionamento utile del *made in Italy* e dei nostri prodotti all'estero. Cito poi le agevolazioni fiscali per la annualità del 2023 a favore del comparto olivicolo

tale comparto, fortemente colpito da questo batterio. Grande assente è la proroga per il credito agricolo. Sono in imminente scadenza le misure straordinarie attivate durante la fase pandemica e questo viene richiesto dalle associazioni di categoria, per dare liquidità agli imprenditori che si trovano col fiato sul collo dei vari creditori. La situazione, infatti, è davvero drammatica. Siamo riusciti a ottenere la proroga per l'acquisto dei beni materiali e immateriali relativi al credito d'imposta 4.0, in quanto la crisi pandemica e il successivo conflitto in Ucraina hanno determinato la fortissima compromissione dell'*iter* di approvvigionamento delle materie prime e questi forti forti ritardi nella consegna dei beni acquistati rischiavano di compromettere il credito maturato. È dunque essenziale essere andati incontro a queste richieste. Abbiamo ottenuto anche la proroga delle misure in tema di occupazione del suolo pubblico per il settore della ristorazione, quindi l'estensione della possibilità di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione, di strutture amovibili in aree di interesse culturale e paesaggistico per gli esercizi pubblici, che dà una boccata d'aria a chi fa ristorazione, continuando ad ammortizzare le gravissime perdite economiche registrate durante la pandemia, che adesso continuano con il caro energia. *In* *extremis* è rientrata la proroga al 30 giugno dello *smart working* per i lavoratori fragili, sia nel pubblico sia nel privato

lavorerà per migliorare quanto di buono già c'è, dando continuità e certezze, perché una strada maestra c'è, quella che sancisce i diritti, che non sono i diritti TV sullo sport del cosiddetto emendamento Lotito che si è riusciti a far stralciare. Mi riferisco ai diritti primari: non si può perdere tempo prezioso in strade secondarie, che risultano essere impraticabili.

La Lega è orgogliosa di aver centrato pienamente alcuni obiettivi della propria azione politica, tra cui mi preme sottolineare la soluzione della questione balneari. Per comprendere quanto fosse importante trovare una soluzione condivisa credo sia sufficiente dare dei numeri. Parliamo di 30.000 imprese nel settore turistico balneare, di cui 7.000 che gestiscono direttamente stabilimenti balneari e circa 23.000 operatori che erogano servizi accessori nell'indotto, quali bar, ristoranti o altri servizi della nautica da diporto. Gli occupati nel settore turistico balneare sono 300.000 e il valore aggiunto del comparto Per noi è sempre stato indispensabile tutelare i nostri imprenditori, tutti i lavoratori coinvolti e difendere il turismo balneare, che una delle voci più importanti del PIL di molte delle Regioni d'Italia. La direttiva Bolkestein, approvata dalla Commissione europea nel 2006 e recepita nel nostro ordinamento nel 2010, chiaramente ispirata ai principi eurounitari di concorrenza e non discriminazione, mira a creare un mercato unico dei servizi incentrato sui pilastri della libertà di circolazione dei servizi e di stabilimento dei prestatori. Si tratta senza dubbio di un testo normativo fondamentale nella misura in cui regola e tutela la prestazione di servizi intracomunitari, dettando norme di armonizzazione, cooperazione amministrativa e semplificazione tali da rendere più agevole l'accesso alle attività dei servizi e il loro esercizio nei Paesi membri. Cionondimeno è stato un testo controverso, che ha avuto un impatto dirompente sul sistema italiano delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ingenerando notevoli problemi interpretativi, che hanno dato vita a un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la compatibilità grazie a tutto con Gian Marco Centinaio Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, era stato avviato un percorso per restituire al nostro Paese sovranità nazionale sulla custodia delle coste attraverso la valorizzazione del bene dato in concessione, in equilibrio con l'ordinamento giuridico interno e unionale, con il fine ultimo di sterilizzare gli effetti distorsivi della direttiva Bolkestein. Purtroppo, però, allora non è stato possibile portare a termine questo percorso e nel novembre del 2021, facendo seguito alle lettere di messa in mora dell'Unione europea, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha riconosciuto l'incompatibilità con l'ordinamento europeo delle proroghe delle concessioni, fissando al 31 dicembre del 2023 il termine ultimo di durata delle stesse. Oggi, preso atto che la questione balneari non è un argomento che rientra nel programma di azione per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, abbiamo proposto una modifica alla legge n. 118 del 2022, con la quale il Governo era intervenuto per evitare che da subito le concessioni fossero considerate abusive e non correre quindi il rischio di andare a gara in assenza di criteri omogenei su tutto il territorio nazionale. Intanto è importante focalizzare la nostra attenzione sul fatto che i giudici della Corte di Lussemburgo nel 2016 hanno definito,

a livello nazionale se la risorsa naturale delle spiagge sia scarsa. Ad oggi nessuna autorità nazionale ha potuto dimostrare oggettivamente che il bene sia scarso. Lo Stato italiano è chiamato quindi a verificare con una mappatura precisa se c'è o se non c'è scarsità della risorsa, facendo anche una ricognizione dettagliata delle aree demaniali già censite come insediamento turistico e ricreativo-balneare, ma non ancora assegnate. Per fare ciò nei giorni scorsi dal MEF è stato istituito il Siconbep, il nuovo sistema informatico per mappare le coste italiane, previsto dall'articolo 2 della legge concorrenza n. 118 del 2022. È indispensabile avere dati oggettivi e non è possibile che l'Italia affidi le sorti di una gestione di un settore così trainante della propria economia a dati forniti da Legambiente. Il Sid, il sistema informativo del demanio marittimo ha iniziato un lavoro di ricognizione e il risultato che emerge è che su 3.347 chilometri totali di costa solo il 43 per cento è concesso, mentre il 57 per cento è. Persino questo dato, però, non risulta significativo, perché a livello nazionale non esiste una norma che stabilisce una percentuale massima di coste che possano essere date in concessione. Le Regioni, infatti, hanno legiferato in modo autonomo sulla percentuale da lasciare libera, che oscilla tra il 60 per cento di Puglia e Sardegna, il 20 per cento dell'Emilia-Romagna, passando per cento del Lazio e il 30 per cento della Calabria. Grazie all'emendamento a nostra prima firma, sarà possibile istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico che coinvolgerà tutti i Ministeri competenti, le Regioni e le associazioni di categoria, con compiti consuntivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Finalmente si definiranno i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale, sia di quello disaggregato a livello regionale, nonché della rilevanza economica transfrontaliera. La proroga di ulteriori dodici mesi è funzionale unicamente all'espletamento di questo importantissimo lavoro. Deve essere chiaro che la Lega, in pieno accordo con la maggioranza di Governo, intende garantire massima osservanza delle direttive europee, ma nel rispetto degli interessi nazionali, che per l'Italia in questo settore sono fondamentali. Gli effetti distorsivi della direttiva Bolkestein devono essere risolti e non si può prescindere dalla fotografia dello stato di fatto delle nostre concessioni. La soluzione trovata va esattamente in questa direzione e permetterà di ascoltare e di coinvolgere le associazioni di categoria. Allo stesso tempo, abbiamo ritenuto necessario anche tutelare i sindaci e gli amministratori locali dall'eccessivo potere discrezionale che era stato loro concesso, in modo da evitare ogni possibile controversia giuridica che li riguardi. Nello scenario attuale, è impensabile che sia un sindaco a poter decidere se e con quali criteri bandire una gara grazie a tutto promessa mantenuta. La politica deve essere fatta di scelte giuste e coraggiose soprattutto per mettere in atto ciò che realmente serve al Paese e con questo provvedimento siamo sicuri di avere iniziato a farlo. cosiddetto milleproroghe poteva essere, come è accaduto varie volte con Governi di diverso colore politico, l'occasione per affrontare una serie di nodi politici, di questioni concrete di interesse per le famiglie e per le imprese lasciati irrisolti dalla legge di bilancio e così poteva essere anche in questa occasione. In realtà, questo non è avvenuto e arriviamo a discutere nell'Aula del Senato un provvedimento rilevante come il decreto milleproroghe in forte ritardo in forte ritardo e non perché le Commissioni competenti si siano impegnate a fondo su nodi di grande portata e di interesse generale, ma perché la maggioranza ed il Governo hanno impiegato il tempo della discussione nelle Commissioni referenti concentrandosi su vicende minori, sicuramente molto importanti per gli interessi particolari toccati dalle scelte fatte, ma sicuramente non strategiche e non riguardanti l'interesse generale del Paese. Ne elenco alcune a beneficio dei colleghi. Abbiamo discusso in Commissione della proroga dei diritti televisivi sul calcio da tre a una proroga che addirittura ha suscitato una levata di scudi dal colle più alto e che quindi il Governo e la maggioranza si sono rimangiati, tant'è che stanno tornando velocemente sui propri passi. alla proroga delle concessioni balneari, di cui ha testé parlato il collega della Lega, il Governo ha deciso che il Paese si deve prendere ancora un anno di tempo per un tema su cui, nella precedente legislatura, il precedente Governo e la precedente maggioranza avevano lavorato intensamente, raggiungendo un compromesso faticoso, con tutti i limiti delle intese tra opzioni molto diverse tra di loro, ma questo compromesso di fatto viene rinviato di un anno con una soluzione che non aiuta gli operatori, perché rimarranno un anno in più in una condizione di incertezza per quanto riguarda le loro attività, e tanto meno aiuta i consumatori e gli utenti rispetto ad una vicenda che invece ha le ha le potenzialità per migliorare i servizi rivolti ai cittadini e agli utenti delle concessioni balneari del nostro Paese. Il rinvio di un anno che non rappresenta certo un bel segnale nei confronti dell'Unione europea su una materia sensibile rispetto alla quale siamo osservati speciali che in altri Paesi ha provocato conseguenze negative. Questa scelta, quindi, a nostro giudizio, giudizio, produrrà delle conseguenze non positive su tutti gli interessi in gioco. Questo è un decreto che ha prorogato altra tematica molto specifica - al 31 marzo la possibilità per i Comuni di aderire allo stralcio delle multe e delle cartelle. abbiamo molto contestato, durante la discussione della legge di bilancio, le dodici norme di condono contenute in quel provvedimento, tra cui in particolare lo stralcio delle cartelle, che da solo costa ai cittadini oltre 1,1 miliardi di euro. All'interno di quella scelta abbiamo criticato ancor di più il fatto che il Governo si faceva bello con i soldi dei Comuni. Il Governo ha poi cambiato orientamento per quanto riguarda le multe e le cartelle di competenza degli enti locali, ma lo ha fatto non prevedendo una compensazione per i Comuni, ma scaricando sui sindaci l'onere della scelta, con il risultato che l'Italia si è mossa a macchia di leopardo. Alcune amministrazioni hanno deciso di stralciare le cartelle di propria competenza e altre, che non avevano questa possibilità, oppure che hanno deciso politicamente in senso diverso, non hanno provveduto allo stralcio. Che cosa fa dunque il Governo? Proroga ulteriormente, di tre mesi, questo scempio della certezza a cui avrebbero diritto i contribuenti, rispetto ad una scelta che è in sé molto criticabile, come abbiamo fatto in sede di discussione della legge di bilancio. Ci si è concentrati su questioni specifiche, su interessi particolari e lobbistici e non si sono affrontati molti temi di interesse generale, che riguardavano milioni di famiglie e milioni di imprese italiane. Questi nodi, che abbiamo ereditato dalla legge di bilancio per sono rimasti del tutto aperti. È rimasto aperto il grande nodo dell'energia, perché le risorse stanziate dalla legge di bilancio finiscono il 31 marzo 2023 e nulla è dato sapere su cosa accadrà dal 1o aprile. Avevamo chiesto di prorogare o comunque di prevedere una fuoriuscita più graduale rispetto al taglio delle accise sulla benzina e sul gasolio: il Governo ha fatto una scelta diversa e nel giro di poche settimane nuovamente di 30 centesimi le accise su benzina e gasolio, con un effetto che ognuno di noi può constatare quotidianamente, andando a a fare benzina. Questo per non parlare del pasticcio che ha provocato lo sciopero degli esercenti, dei benzinai, in ragione delle scelte assurde che il Governo ha assunto su questa materia. Avevamo chiesto di prorogare il taglio dell'IVA al 5 per cento sul teleriscaldamento, che è una realtà che riguarda centinaia di migliaia di famiglie italiane, in Comuni grandi e piccoli: penso a Milano, a Torino, a Bergamo o a Brescia, ovvero a realtà in cui il teleriscaldamento è una modalità molto diffusa e ormai generalizzata di riscaldamento degli edifici. Il Governo ha fatto una scelta importante per il primo trimestre, ne avevamo chiesto la proroga, ma ci è stato detto di no. Torneremo alla carica, naturalmente, perché perché ci siamo battuti molto in passato per questa scelta e riteniamo sia necessaria una parità di trattamento fiscale, rispetto al taglio dell'IVA che è stato effettuato sul gas, ma il Governo su questo e su altri temi energetici no, così come ha detto di no all'emendamento per prorogare al 2024 il termine per la fine della tutela del prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia. Il Governo ci ha detto di no su temi importanti che riguardano il lavoro e la previdenza. Opzione donna è uscita fortemente indebolita dalla legge di bilancio, con penalizzazioni del tutto ingiustificate, rispetto a tante lavoratrici che in passato avevano potuto usufruire di questo canale accelerato di ingresso nel sistema pensionistico. Avevamo chiesto di ripristinare i criteri in vigore fino al 31 dicembre 2022, ma il Governo ci ha detto di no. Sempre parlando di lavoro, il

Ci siamo impegnati sulla sanità: in questo caso alcuni passi avanti sono stati registrati e ne diamo atto al Governo. Sono stati accolti emendamenti su cui ci eravamo impegnati: penso al tema della stabilizzazione dei medici e degli specializzandi in servizio durante il Covid, penso alla tematica dei medici di medicina generale, dei pediatri e del personale di ricerca, alle professioni sanitarie e alla formazione del personale sanitario. Naturalmente ereditiamo dalla legge di bilancio il nodo di un sottofinanziamento del Fondo sanitario nazionale che si ripercuoterà su tutte le Regioni italiane, a partire da quelle che negli anni drammatici del Covid hanno difeso la sanità pubblica, hanno difeso i lavoratori e le lavoratrici del Servizio sanitario nazionale.

parlando degli enti locali e delle soluzioni parziali o insufficienti che sono state date alle istanze dei Comuni e degli enti di Area vasta che erano rimaste irrisolte con la legge di bilancio. Per tutti questi motivi, signor Presidente, il nostro giudizio su questo decreto-legge è critico. Riconosciamo alla maggioranza e al Governo di aver accolto numerosi emendamenti dell'opposizione e questo lo dobbiamo dire per onestà intellettuale. Tuttavia, Presidente, serviva e serve ben altro per affrontare i nodi più urgenti a cui devono far fronte le famiglie e le imprese italiane.

oggi si discute un decreto-legge il cui contenuto si traduce nel prorogare o differire termini su disposizioni che, in alcuni casi, questo Governo ha confermato valide; in altri, invece, vuole più tempo. Vuole più tempo per una valutazione di merito e, quindi, per attuare misure che possono incidere in maniera più efficace su interessi rilevanti, che toccano famiglie, lavoratori e settori produttivi. Prima di entrare nel merito di alcune disposizioni, desidero sottolineare l'impegno profuso dalle Commissioni 1a e 5a riunite al Senato nel concludere la trattazione di un provvedimento così ampio e trasversale. Fondamentale è stato il lavoro svolto dal Governo, che ringrazio: finalmente oggi alla guida di questa grande Nazione c'è un Governo voluto dalla maggioranza degli italiani. un Governo che dimostra di lavorare incessantemente per costruire una Nazione più dinamica, competitiva e al passo con le sfide del nostro tempo, nonostante i continui proclami apocalittici, smentiti puntualmente nei fatti, di chi dimentica o non si rassegna al fatto di essere stato bocciato alle urne dai cittadini italiani che hanno scelto e che continuano anche oggi a scegliere in modo democratico - e sottolineo democratico - da chi vogliono essere rappresentati.

che ha dovuto curare i contatti con tutti i Ministeri, e a tutta la maggioranza per i risultati raggiunti. Tra le misure previste nel decreto-legge,

d'Italia, integrativi rispetto alle misure già previste e riguardanti scuola, università, sanità ed enti locali, emendamenti approvati nelle Commissioni riunite e frutto di un grande lavoro e di un'ampia convergenza da parte dei colleghi della maggioranza. Con l'approvazione dell'emendamento che prevede un corso concorso con selezione e prova finale per la qualifica di dirigenti scolastici si chiude oggi un cerchio, mettendo la parola fine su uno dei concorsi più discussi degli ultimi anni, quello del 2017. Quindi, con un decreto ministeriale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di questo provvedimento, si definiscono le modalità e lo svolgimento È riservato ai soggetti che abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta, della prova orale ovvero abbiano superato sia la prova scritta o la prova orale, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare. Voglio ribadire - e lo ribadisco a chiare lettere - che Fratelli d'Italia non propone una sanatoria: nessun canale preferenziale. Noi non vogliamo abbonare o condonare nulla a nessuno. Basta con attacchi critici - basta! - per celare solo ed esclusivamente la verità dei fatti. Nell'ottica del merito, in cui crediamo fermamente, permettiamo invece a chi è stato eliminato da una procedura ingiusta di riprendere il suo percorso concorsuale, conciliando così due valori fondamentali, due fari per Fratelli d'Italia: il merito e la giustizia. Merito e giustizia per chi ogni giorno continua a servire lo Stato, educando le generazioni del futuro e continuando, nonostante tutto, a infondere nei nostri studenti la fiducia nelle istituzioni. Un piccolo passo si è fatto per gli idonei del concorso straordinario *bis*, con l'approvazione dell'emendamento che prevede sia la proroga di un anno per l'assunzione dei docenti vincitori, considerati anche i ritardi per alcune classi di concorso che di fatto hanno impedito di effettuare le nomine in tempo utile, sia la possibilità di scorrimento della graduatoria nel caso di eventuali rinunce. Certo è che il nostro lavoro non si ferma qui. Tanti ancora sono i *dossier* aperti, sui quali continueremo a impegnarci per restituire dignità e certezza a questa grande istituzione, che in tutti questi anni è stata abbandonata da tempo, da chi era precedentemente al Governo, che nulla ha fatto e che improvvisamente si sveglia e solleva inutili e sterili polemiche. Importanti sono gli emendamenti di Fratelli d'Italia sull'università. Attraverso essi si è consentito di ultimare gli oltre 400 corsi formativi ancora attivi del percorso vecchio ordinamento AFAM, rallentato a causa della pandemia Covid. Così si è riusciti a garantire che i diplomandi acquisiscano un titolo che in effetti altrimenti non sarebbe spendibile a causa della mancata equipollenza. Altro emendamento importante è quello che permette agli atenei una migliore programmazione, anche in funzione della semplice considerazione dei differenziali di costo del personale, prevedendo l'estensione fino al 2026 delle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato. Il lavoro sul decreto milleproroghe è stato molto complesso anche nel settore sanità. Importante è l'emendamento che consente ai medici di medicina generale e ai pediatri, entrambi convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, la possibilità di andare in settantadue anni e non a settanta. Quindi da oggi il Servizio sanitario avrà uno strumento in più per contrastare la carenza di personale che sta colpendo ogni Regione italiana. siamo riusciti a far rientrare anche i dipendenti amministrativi delle strutture sanitarie nei piani di stabilizzazione del personale, aiutando quei lavoratori che nel periodo della pandemia sono stati importanti quanto i medici.

affari costituzionali e bilancio, e grazie al grande lavoro di supporto da parte del ministro Ciriani e alla serietà e sensibilità del Governo su un tema estremamente delicato che riguarda i lavoratori fragili - attraverso la copertura finanziaria di ben 16 milioni fornita, oltre che dal Ministero del lavoro, anche dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione e del merito - si è riusciti a prorogare di tre mesi lo *smart working* per i lavoratori fragili e per la sostituzione di tale personale. Questo è un vero successo di tutti. Rilevante è tutto il lavoro che abbiamo fatto. conclusione, Presidente, con questo decreto-legge è stato fatto, come ho già detto, un lavoro importante, sinergico e incisivo su tanti temi. Ciò che mi preme oggi sottolineare è che finalmente è ritornato nelle Commissioni il dibattito parlamentare il rispetto delle opposizioni. Si è ristabilito il corretto confronto istituzionale attraverso un costante dialogo con il Governo che non è mai mancato e che ha dimostrato e continua ogni giorno a dimostrare di essere all'altezza del momento complicato che stiamo vivendo e di avere un unico obiettivo: dare risposte agli italiani e ai molti settori in crisi e in difficoltà. Signor Presidente, le catastrofi preannunciate e le innumerevoli critiche strumentali lasciamole a chi vuole nascondere il proprio fallimento dimostrato in tutti questi anni.

della proposta. Spiegai all'allora presidente Monti, tuttora nostro collega come senatore a vita, reduce fresco dall'esperienza decennale di commissario europeo, che per l'Italia le spiagge erano una particolarità, perché due terzi d'Europa non le usa per ragioni climatiche; le usa il giorno di Ferragosto. Il Sud della Francia, l'Italia, la Spagna, la Grecia e altri pochi Paesi hanno nelle spiagge una risorsa per il turismo e per l'economia; quindi, una considerazione speciale ci doveva essere. In più, noi diciamo da tempo che la direttiva Bolkestein non andrebbe applicata perché riguarda una concorrenza relativa ai servizi, e qui siamo di fronte a beni. Lo stesso Bolkestein - lo ricorderà anche il presidente Centinaio - venne in Italia anni fa a un convegno nell'Aula dei Gruppi parlamentari spiegando che la sua famosa direttiva non riguardava quel settore. Ma Bolkestein non è più commissario europeo e la sua interpretazione autentica fa parte del dibattito, ma non risolve la questione. Dopodiché, siamo andati avanti con la scadenza del 2020; lei, che presiede oggi l'Assemblea, era Ministro dell'agricoltura con delega anche al turismo;

Ci fu una condivisione ampia, anche da parte di Gruppi che oggi sono critici, non voglio rivendicare solo per Forza Italia con Gasparri e Mallegni o per la Lega con il ministro Centinaio e altri. Dopodiché, c'è stata la sentenza del del Consiglio di Stato, basata a mio avviso - lo dico nel massimo rispetto del Consiglio di Stato - su premesse false. In quella sentenza ci sono pezzi quasi di volantini o di editti

le mareggiate. Chissà se il selettore del candidato Soumahoro ha consapevolezza - mi riferisco a colleghi di altri Gruppi - che anche durante questa stagione il il mare spazza via aziende che sono fragili. C'è l'erosione delle coste, ci sono tanti problemi. Quindi uno ha lo stabilimento, ma poi non ce l'ha più; ha una spiaggia ma poi non ce l'ha più.

ha voluto fare una legge sulla concorrenza, abbiamo cercato di convincerlo che era sbagliato e devo dire che anche il Governo Draghi ha cominciato a inguaiarsi quando ha litigato con alcune categorie italiane. Se avesse ascoltato meno Giavazzi, forse Draghi sarebbe arrivato alla fine della legislatura, ma il "giavazzismo" è una malattia infantile o senile del liberismo. Si è voluta fare una norma, abbiamo introdotto il termine del 2023

proroga dal 2024 al 2025. Abbiamo chiesto di fare un tavolo per discutere con le categorie. Il Governo ha ascoltato le categorie e ha espresso parere positivo su questi emendamenti. I relatori ne hanno aggiunti altri due che riguardano altri aspetti tecnici: il blocco ai Comuni per quanto riguarda le gare

e domani volessi farlo, potrei mettermi in coda e partecipare all'assegnazione di aree non ancora assegnate. Vogliamo anche le spiagge libere, ma queste non sono le spiagge abbandonate: sono le spiagge dove c'è il bagnino e la sicurezza. I Comuni le devono fare e le devono tenere pulite. Quindi quelli che fanno la propaganda alle spiagge libere, Le spiagge libere ci devono essere, ma devono essere accessibili, pulite e vigilate, in modo che chi voglia andare alla spiaggia libera non vada nel deserto o nella discarica. Potrei aggiungere altre cose. Sono contento che i nostri emendamenti siano stati approvati in Commissione da tutto il centrodestra. Sono certo che anche i colleghi che hanno un po' nicchiato siano d'accordo. Mi auguro che la smettano di dire bugie e che il Consiglio di Stato si ravveda

dialettica e un ottimo dialogo anche con le opposizioni e fra i Gruppi di maggioranza. È stato il primo provvedimento così corposo che abbiamo affrontato in Commissione con questo nuovo Governo, quindi è stato un bel banco di prova. È un provvedimento molto tecnico e questo ha facilitato anche i rapporti con la minoranza, la quale ha dato assieme a noi un importante contributo su diversi aspetti che sono stati toccati nei giorni di lavoro in Commissione. Si tratta di un provvedimento molto eterogeneo, quindi non mi soffermerò su tanti temi importanti, perché l'hanno fatto o lo faranno altri colleghi. Ognuno di noi, così come gli altri Gruppi di maggioranza, ha cercato di dare il proprio apporto, in base ovviamente alle proprie competenze e anche al proprio ruolo nelle varie Commissioni. Ricordo però, su tutti, alcuni emendamenti molto importanti sul tema della disabilità, con la proroga della legge

abbiamo collaborato per l'approvazione anche di emendamenti delle minoranze. Penso alla proroga della ricetta elettronica, che è un emendamento di assoluto buonsenso, o alla continuazione del finanziamento del Piano oncologico nazionale, che è molto importante. Il Gruppo parlerà poi dell'importante problema della carenza dei medici di medicina generale e anche di quello delle liste d'attesa. Anche su questi temi principali siamo riusciti a dare il nostro piccolo contributo.

Parliamo di una norma importante, che prevede lo scorrimento delle graduatorie per il personale della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, e in particolare il ruolo degli ispettori di Polizia, che da tempo è segnato da gravi scoperture rispetto alla dotazione organica, stabilita dalla normativa vigente. Oltretutto, ad aggravare questo problema c'è anche il forte incremento dell'età media del personale, quindi nei prossimi anni il grande *gap* già esistente potrà peggiorare proprio per questo motivo. Abbiamo Abbiamo dunque previsto un incremento del ruolo del direttivo, di 637 unità, e un'ulteriore alimentazione della qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato per 1.735 unità e 1.141 posti posti di vice ispettore. Sempre riguardo alle Forze dell'ordine, è previsto un importante intervento di semplificazione per le assunzioni e per i corsi di formazione per le Forze di polizia e lo scorrimento delle graduatorie anche della Polizia penitenziaria. Questo è importante anche in vista degli eventi per cui sarà necessario il supporto di tutte le nostre Forze di polizia, e non solo, per il Giubileo del 2025 e per le Olimpiadi invernali del 2026. Da ultimo, abbiamo affrontato diverse tematiche relative agli enti locali per quanto riguarda il PNRR. Vi è stato un importante confronto tra di noi e col Governo. Così dovrebbero svolgersi, secondo me, i lavori della Commissione. Ciò è servito, infatti, anche per dare spunti al nuovo decreto PNRR, dal momento che non abbiamo potuto risolvere qui tutti i problemi collegati ai bandi. Spero che questo modo di lavorare, in cui si entra tanto nel merito si riesce a discutere bene anche con le minoranze, dando atto del lavoro che ognuno di noi cerca di fare per il bene della nostra gente e del nostro territorio, possa essere portato ad esempio anche nei prossimi provvedimenti, un po' più politici e meno tecnici.

una strategia di economia finanziaria e di sviluppo del Paese che ci avrebbero portato a investire su quei pezzi di PIL che sono andati così bene in questo anno e mezzo, in cui abbiamo avuto un rimbalzo del 6,6 per cento, per portarci a crescere anche nei prossimi anni.

signor Presidente, sono una ragazza di periferia e vado al mare a Ostia, dove ho la cabina da sempre, quindi non vado in spiagge *radical chic*; eppure, sulla questione dei balneari, piuttosto che sturare le orecchie all'Europa temo le sturino a noi, per cui abbiamo un problema serio. Intendo dire che chi fa balneazione in Italia vuole avere delle certezze,

Come Partito Democratico - e cito gli emendamenti a firma Zampa, Lorenzin, Nicita, Manca e tanti altri - abbiamo cercato di portare a casa, diciamo così, le proroghe che ci permettono quanto meno di mantenere una dinamica dell'occupazione e della stabilizzazione dei precari, ma anche di intervenire sui pensionamenti, sull'assenza di personale specialistico, sui medici di medicina generale e sui pediatri di libera scelta. Purtroppo è rimasto fuori il personale di ricerca (come se la ricerca non fosse un elemento fondamentale dello sviluppo e dell'assistenza del nostro Paese), come pure altri comparti, perché non c'è stata la capacità di andare oltre, oltre, permettendoci di raggiungere un obiettivo, quanto meno nell'attesa di una proposta di riforma complessiva sul personale sanitario italiano, tale da renderlo più attrattivo, evitando certi esodi e riuscendo a garantire il servizio. Lo dico perché abbiamo ancora questo problema, che non è risolto e che vedremo crescere nei prossimi mesi. Faccio un appello su due emendamenti che abbiamo ripresentato: uno sul *bonus* psicologico

abbiamo perso un'occasione per dare una risposta a chi ne ha veramente tanto bisogno e spero che il Governo ci permetta di affrontare di nuovo questo tema in un altro tavolo.

ma il lavoro che abbiamo svolto insieme lo ha ulteriormente arricchito, anche con un importante contributo in termini di emendamenti dei senatori del Gruppo Forza Italia, che sono stati approvati nel corso dell'esame delle Commissioni riunite.

con il *record* del Comune di Moncenisio, con soli 30 residenti. Per questo sono soddisfatto che le nostre proposte a favore dei piccoli Comuni siano state accolte. Sappiamo che in generale la carica di sindaco origina grandissime difficoltà e responsabilità, ma nei piccoli Comuni a volte bisogna essere eroi per svolgere il ruolo del primo cittadino. A volte, si stenta a trovare tra la popolazione chi si vuole sobbarcare a questo gravoso compito e, quando si trova, si rischia che non ci sia l'affluenza necessaria per eleggerlo. Ecco perché è importante l'accoglimento della mia proposta di estendere anche per l'anno 2023 la norma per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni fino a 15.000 abitanti, ove ammessa e votata una sola lista, che siano eletti tutti i candidati, compreso il sindaco, purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore a 50 e di votanti non inferiore a 40. Inoltre, per la determinazione del numero di elettori iscritti nelle liste elettorali, non si terrà conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e quindi anche per l'anno 2023 sarà più semplice per i piccoli Comuni eleggere un sindaco e un Consiglio comunale. Considerato il calo della partecipazione al voto, che purtroppo abbiamo visto anche ieri, spero che questa norma diventi definitiva e non rimanga solo una proroga, così come spero che diventi legge la proposta di Forza Italia, a mia prima firma, di eliminare i limiti di mandati per i sindaci dei piccoli Comuni. La seconda proposta che riguarda i Comuni affronta un altro grande problema, quello della carenza dei segretari comunali. L'emendamento è stato recepito dal Governo e devo ringraziare il ministro Zangrillo e il ministro Piantedosi per il grande lavoro svolto per rendere efficace la norma. Sappiamo che la carenza dei segretari fa sì che la maggior parte dei piccoli Comuni ne possa usufruire per poche ore alla settimana, con casi estremi in cui un segretario comunale è a scavalco su 14 Comuni. In un momento così importante per il Paese, in cui sappiamo che dobbiamo sfruttare al meglio le risorse a nostra disposizione come quelle del PNRR, i piccoli Comuni sono praticamente tagliati fuori, privi della necessaria consulenza tecnico-giuridica che un segretario comunale può fornire. Un passo avanti per risolvere il problema è stato fatto quindi grazie a questo emendamento, che è stato assorbito dal Governo e che prevede, al fine di supportare proprio l'attuazione del PNRR per la durata del medesimo piano, che il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera su richiesta del sindaco possa assumere la titolarità anche in sedi corrispondenti alla fascia professionale alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino a 5.000 abitanti e questo per dodici mesi rinnovabili fino a Certo, i piccoli Comuni hanno anche carenza di risorse per pagare i segretari comunali, ma questo problema pure è in fase di soluzione, stante che il ministro Zangrillo ha già stanziato nella legge di bilancio 30 milioni di euro, destinati ai Comuni per questa finalità. Nel campo del superbonus è importante che sia stata accolta, anche se come raccomandazione, la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per gli interventi effettuati sugli immobili di proprietà

rimane ancora il problema dei crediti incagliati. *(Applausi)*. Le imprese del mondo dell'edilizia sono in sofferenza ed è evidente che la soluzione del prestito garantito Sace non sia risolutiva per tutte le situazioni. Dei molti altri temi trattati da Forza Italia parleranno i miei colleghi. Dunque, è un ottimo lavoro quello del Governo sul milleproroghe, arricchito dall'esame in Senato. Nonostante questo, purtroppo, continuo a sentire critiche provenienti dall'opposizione sull'operato del Governo e della maggioranza, un'opposizione che pensa sempre di avere la verità in tasca. I cittadini lombardi e laziali, però, ieri hanno dato fiducia al centrodestra in misura maggiore che alle scorse politiche. un evidente segno di gradimento anche dell'operato del Governo, ma anche su questo fatto ho sentito esponenti dell'opposizione dire che si trattava di elezioni locali e che quindi non contano. Si dice che chi vive di illusioni vive meglio: rimanete pure a crogiolarvi nelle vostre illusioni, mentre il centrodestra unito, coeso e vincente affronta la realtà e risolve i problemi dei cittadini e delle imprese italiane.

Il decreto milleproroghe viene emanato a fine anno per posticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni normative o per prevedere deroghe alle disposizioni disposizioni normative in vigore. Esso è sicuramente un provvedimento che, in un momento di crisi economica come quella in cui versa il nostro Paese, possiamo considerare come un'ancora di salvezza per molti e un sospiro di d'Azione anche nel provvedimento in esame ha cercato di portare le istanze raccolte nei territori e di renderle effettive, con la consapevolezza che le criticità del momento interferiscono con molte attività sociali, culturali, imprenditoriali e sulla sanità. Anche le proroghe possono contribuire al mantenimento del benessere sociale ed economico. Entrando nel merito del provvedimento o, per meglio dire, delle modifiche apportate al decreto-legge, vorrei citarne alcune,

d'Azioneavevamo proposto un emendamento che desse questa possibilità a tutti i medici, proprio per coprire la carenza di personale. Ci sono, inoltre, l'estensione delle ore di libera professione per infermieri e ostetrici, il *benchmark* per la determinazione del fabbisogno sanitario *standard* e la quota premiale del Fondo sanitario nazionale 2023. Inoltre, è prevista una proroga per i fondi destinati al piano oncologico nazionale. Altro tema importante per la sanità è il rinvio del *payback* sanitario al 30 aprile. Si tratta di un tema importante, per cui va necessariamente trovata una soluzione e di cui voglio ricordare la genesi. Nel 2015, epoca di emergenza finanziaria causata dal pesante disavanzo in cui versavano quasi tutte le Regioni, che infatti erano in piano di rientro, furono decisi dei tagli lineari. La spesa del Servizio sanitario nazionale per i dispositivi medici rappresentava all'epoca il 5,2 per cento dell'intera spesa sanitaria e dunque fu fissato un tetto alla spesa del settore, pari al 4,4 Considerando che tale tetto sarebbe stato superato, fu previsto anche per i dispositivi medici lo strumento del *payback*. Il meccanismo del *payback* prevede che, partendo dal tetto nazionale al 4,4 per cento, mai modificato, il Ministero della salute ogni anno avrebbe dovuto definire il tetto per ciascuna Regione, in quanto ogni Regione ha un proprio tetto, che dipende dalla quantità di privato convenzionato operante sul territorio regionale. La quota di spesa che eccede eccede il tetto dev'essere rimborsata in parte dalla Regione stessa all'interno del proprio bilancio, in parte dalle imprese del settore. Per il 2015 era previsto il 40 per cento a carico delle imprese, dal 2016 in poi il 50 Dunque, sulla base di tale meccanismo, la Regione acquista e, successivamente, se al termine dell'annualità risulta lo sforamento del tetto, chiede ai fornitori di restituire la metà della spesa che eccede il tetto. Questo provvedimento è stato emanato nel 2015 e purtroppo il decreto-legge aiuti-*bis* ha confermato il *payback* sui dispositivi sui dispositivi medici: ultimo regalo del ministro Speranza. Il settore dei dispositivi medici in Italia genera un mercato che vale 16,2 miliardi di euro, tra *export* e mercato interno, e conta 4.546 aziende, che occupano 112.534 dipendenti. Si tratta di un tessuto industriale molto eterogeneo, altamente innovativo e specializzato. Con l'applicazione di questa normativa si mettono a rischio tale tessuto produttivo - che si pone come settore cruciale per la sanità ed è inoltre un'eccellenza del Paese con il pericolo di perdere quest'eccellenza - le forniture di prodotti e di apparecchi salvavita per gli ospedali. Il rinvio del *payback* al 30 aprile dev'essere accompagnato da un tavolo tecnico di confronto, come richiesto dal mio ordine del giorno approvato in Commissione, per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. Un altro settore su cui bisognerà porre attenzione è quello dei distributori farmaceutici. I sempre maggiori costi e minori ricavi hanno aggravato la situazione; la distribuzione intermedia farmaceutica è riconosciuta quale servizio pubblico essenziale e come indispensabile anello di collegamento fra la produzione industriale e la dispensazione finale al pubblico, con particolare attenzione alle esigenze di tutela della salute e della qualità della vita della collettività. Uscendo dal tema della sanità ed entrando nel mondo del lavoro, esprimo soddisfazione per l'emendamento che proroga per ulteriori tre mesi nel settore privato, fino sia ai lavoratori fragili, sia a quelli con figli fino ai quattordici anni, così come per l'emendamento che prevede, per i contratti di somministrazione a tempo determinato, la possibilità d'impiego del lavoratore in missione per periodi superiori a anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato. L'efficacia di tale previsione è prorogata al 31 giugno 2025. Il Fondo nuove competenze è prorogato per il 2023.

subentro del nuovo concessionario. L'autostrada del Brennero rappresenta un presidio indispensabile per lo sviluppo e il protagonismo delle nostre comunità ed è un asse europeo strategico fondamentale per tutto il Paese. In questa direzione va l'emendamento che intende prorogare il termine per il versamento dell'acconto per il subentro del nuovo concessionario dell'autostrada A22, relativo all'anno 2022, anziché, come previsto dalla disposizione, al 30 aprile 2023. La proroga è necessaria per consentire al concessionario di non perdere l'affidamento nel periodo in cui viene prorogata la procedura di finanza di progetto. La Lega dimostra ancora una volta concretezza e attenzione alle esigenze dei cittadini e dei territori. *(Applausi)*.

si può parlare da opposizione e si possono esprimere le proprie convinzioni anche se due giorni prima si sono perse le elezioni. *(Applausi)*. Non è un argomento dire che si ha una critica o la verità in tasca e che quella verità

Inoltre, visto che mi è stato fatto omaggio del calendario del Senato del 2023, invito la maggioranza, in particolare Fratelli d'Italia, a scegliere una qualunque data di questo calendario (la sceglieranno loro), passata la quale si potrà finalmente dire che c'è una responsabilità nelle scelte di questo Governo e non soltanto di quelli precedenti. Ciò detto, passando la parola «proroga» secondo l'Enciclopedia Treccani è la prosecuzione consentita dal rinvio di una scadenza: la maggior parte delle cose che questa maggioranza ha deciso di prorogare le aveva decise un altro Governo, sempre per dare un senso alla discontinuità. Noi ovviamente abbiamo approvato alcune cose che facevano parte delle scelte precedenti e mi riferisco in particolare

hanno richiamato il Governo rispetto ad alcuni ritardi, ma anche ad alcune contraddizioni. Un paio di emendamenti, di cui mi onoro

valore al lavoro che ha fatto la Commissione, dall'altra, ci dà la fotografia di un Governo in molti casi impreparato, in diversi casi confuso e contraddittorio, in alcuni casi privo di una linea univoca e in altri casi ancora capace di un capriccioso no, senza spiegarne in dettaglio le ragioni. Ora, tra gli emendamenti che sottolineiamo, ci sono quelli che riguardano i termini della stabilizzazione per il comparto sanitario, ma qui ne ripresentiamo uno, perché uno dei problemi di questi famosi milleproroghe è che spesso prendiamo decisioni

hanno svolto un lavoro prezioso. Nel PNRR abbiamo un quantitativo importante dedicato alla telemedicina e alla digitalizzazione del comparto sanitario, ma poi l'assistente informatico, che ha lavorato e che abbiamo chiamato

di altri professionisti non sanitari che pure sono ricompresi nel decreto, quindi si crea una discriminazione. Ugualmente, si crea una discriminazione per quanto riguarda le giuste risorse trovate per

è stato possibile farlo soltanto per i dipendenti del comparto privato, perché non comporta oneri. Siccome poi dopo si sono trovati degli oneri giustamente e con nostra soddisfazione - per la parte fragile, anche qui recuperando la parte di un emendamento a firma Camusso, ci chiediamo per quale motivo non sia stato possibile estenderlo anche ai dipendenti del settore pubblico. delle misure che dobbiamo portare a sistema. Quello che manca, da parte del Governo, è una visione delle misure che possano essere portate a sistema. La questione del lavoro agile o dello *smart working* non era semplicemente legata a un'eccezionalità: è la sfida dell'organizzazione

con maggior forza e maggiori risorse, ma che non ha trovato sufficiente attenzione. Abbiamo provato a introdurre misure che riguardassero, per esempio, casi specifici territoriali, sui quali abbiamo avuto un diniego. Mi riferisco al mancato incremento dei pedaggi per quanto riguarda l'attraversamento del ponte Morandi, così come ad altre questioni che hanno riguardato vicende territoriali. Mi permetta di chiudere su un punto, Presidente: la questione dei balneari. Qui ho sentito alcune affermazioni che in punto di diritto sono veramente molto deboli, secondo le quali il concetto della direttiva Bolkestein, quindi della concorrenza tra servizi a livello europeo, dipenderebbe dal concetto di scarsità. Attenzione su questo. Il concetto di scarsità fa riferimento all'idea che debba esserci o meno una gara, è vero; ma il concetto di scarsità è un concetto economico e non semplicemente di natura fisica, per cui il fatto stesso che ci sia una domanda in eccesso rispetto all'offerta

facilitare o meno determinate categorie, ma di inserirle in un contesto economico nel quale il valore della concorrenza si riferisce anche a potenziali

difficoltà rispetto allo sviluppo di un mercato; non c'è una riforma. Andiamo verso il rischio di sanzione, e questa è una di quelle proroghe che non avremmo voluto vedere in questo provvedimento.

a Milano si dice «fa ballà l'oeucc» per dire: fa' bene attenzione a quello che fai. Come sapete, ieri e l'altro ieri la stragrande maggioranza degli elettori votanti lombardi e laziali lo ha fatto! Pertanto, ciò vuol dire che gli sforzi che sono stati sin qui fatti, in questi pochi mesi di Governo, dettati dalla concretezza del possibile, sono stati giustamente recepiti. modo, il nostro plauso non scontato al provvedimento in conversione è dovuto soprattutto che, in qualche misura, data la relatività delle risorse disponibili e la consistenza delle problematiche in trattazione, anche in sanità, sono stati previsti importanti interventi che, se daranno gli esiti sperati, ci faranno convintamente proseguire nel percorso finalizzato a dotare il sistema di ciò di cui necessita. Altro che sanità terminale!

e l'altro sul rafforzamento della medicina territoriale, che ci proietteranno nel futuro. Tutto questo anche grazie all'approvazione degli emendamenti che abbiamo proposto e sostenuto, con risorse, come dicevo, senz'altro inadeguate rispetto ai fabbisogni,

dal nostro punto di vista, vede un cambio di passo al fine di valorizzare le potenzialità del sistema per rispondere con sempre maggiore tempestività e appropriatezza alle necessità di prevenzione, di diagnosi precoce e cura, e non solo in oncologia. Le maggiori risorse a sostegno delle misure per il recupero dei tempi di attesa ci fanno auspicare che, entro tempi ragionevoli, il problema sia un ricordo del passato, almeno nelle dimensioni attuali. Sono stati infatti prorogati gli strumenti a disposizione delle Regioni per normalizzare i tempi di esecuzione delle prestazioni, non solo attraverso il finanziamento dell'impegno da parte delle strutture pubbliche, ma anche consentendo di acquistare dal privato, a domanda, le prestazioni su cui si scontano i maggiori ritardi. Il tutto mediante due azioni sinergiche: l'utilizzo dei fondi non spesi per il riequilibrio 2022 e la possibilità di arrivare fino allo 0,3 per cento del livello del Fondo sanitario nazionale 2023, equivalente a circa 400 milioni. Tale doppia azione, unita alle norme di maggiore flessibilità nel reclutamento e nella valorizzazione delle risorse umane disponibili, introdotte in chiave emendativa con un percorso partecipato e condiviso financo con le opposizioni, ci si augura che garantisca in modo rapido il recupero dei ritardi sin qui maturati. Venendo incontro alle necessità e alle richieste dei professionisti, sarà *medio tempore* consentito, su base volontaria, di differire il collocamento a riposo fino al settantaduesimo anno di età. Sarà consentita la possibilità di prorogare, per le strutture del Servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa, la possibilità di assumere gli specializzandi e l'opportunità di esercitare temporaneamente nel territorio nazionale le qualifiche professionali sanitarie e la qualifica di operatore sociosanitario in deroga alla disciplina ordinaria per il loro riconoscimento. È stata infine prorogata ed ampliata la possibilità per gli infermieri e i restanti operatori delle professioni sanitarie del comparto di svolgere la libera professione, seppure nei limiti delle otto ore settimanali. Questo è possibile. Signor Presidente, come hanno ben argomentato i colleghi del mio Gruppo intervenuti prima di me, il provvedimento in discussione, a nostro giudizio, ha dei difetti molto importanti: contiene degli esercizi di liberalismo immaginario; contiene una difesa miope di posizioni corporative; è caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi spirito riformatore. Sembra poi che ci sia la volontà da parte della maggioranza di difenderlo in una maniera a nostro avviso sbagliata, cioè con l'idea che quella del Governo non sia un'attività concreta, consistente nel risolvere i problemi del presente, ma un'attività retorica, consistente nel fare l'opposizione al passato. Questo, secondo noi, è un limite molto forte dell'azione del Governo e in questo provvedimento lo si avverte in maniera particolare. grossissimi difetti, che non potevo non citare molto rapidamente, riteniamo anche che ci sia qualche pregio che va messo correttamente in evidenza. Sono stato al centro di uno di questi pregi e ho incontrato, per portare a casa un risultato importante e di giustizia, la collaborazione del presidente della Commissione, senatore Balboni, e di tutti i Gruppi. Mi riferisco all'emendamento che ha permesso di aprire una nuova finestra temporale di quattro mesi per i parenti delle vittime di eccidi, stragi e deportazioni compiute dal nazifascismo nel nostro Paese, che non hanno fatto in tempo ad avviare le azioni civili di richiesta di risarcimento durante la precedente finestra temporale, quella apertasi nel mese di aprile e chiusasi alla fine del mese di novembre. Forniamo così a persone che hanno subito sofferenze grandissime un'opportunità importante

al ministro Giorgetti, al quale ho già scritto una lettera. Siamo in ritardo di quattro mesi per l'emanazione del decreto ministeriale che deve indicare la procedura da seguire per avere i risarcimenti da parte di coloro che hanno già sentenze definitive e che, quindi, vantano già un diritto ad essere risarciti. Se il Ministero dell'economia e delle queste persone non possono vedere riconosciuto un diritto che, a questo punto, essendo le sentenze definitive, è scolpito nella pietra. Questa inadempienza è molto ingiusta. Pertanto, mi auguro che lo stesso atteggiamento unanime che c'è stato nel riaprire la finestra temporale ci sia anche nel premere sul MEF affinché

di provvedimenti già assunti dal precedente Governo e che non dia la traccia dell'azione innovativa della maggioranza di centrodestra. Intanto, credo che ieri essi siano stati smentiti clamorosamente dagli elettori. Il successo oltremodo importante, che è venuto dalle urne nelle regioni Lombardia e Lazio, dimostra, invece, che questa azione di governo viene percepita come assolutamente concreta, assolutamente efficace ed assolutamente in grado di venire incontro alle esigenze della popolazione. E la gente ce ne dà atto con lo strumento della democrazia. Non è una polemica, è una constatazione. Noi siamo, oggettivamente, un Governo che è espressione di volontà popolare, che continua ad avere consenso popolare. E vivaddio, perché forse per dieci anni questo non era accaduto. *(Applausi)*. Questo provvedimento, quindi, non è una semplice proroga termini, ma è il corollario di un'azione, iniziata con una serie di provvedimenti dal Governo Meloni, e che ha avuto naturalmente il suo apice con la legge di bilancio dello scorso fine anno; legge di bilancio, lo ricordo, condizionata dall'attuale momento economico e politico, a causa del quale buona parte delle risorse disponibili sono state messe

poter intervenire economicamente in questo provvedimento. Pur non di meno, si è cercato, come è stato richiamato da più colleghi della maggioranza negli interventi che mi hanno preceduto, di venire incontro a diverse esigenze, anche dal punto di vista ordinamentale e comunque di efficienza del sistema complessivo della pubblica amministrazione. Mi riferisco, in particolare, alle norme

si è stabilita la possibilità di una stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale nel prossimo triennio a carico delle Regioni, cercando, da un lato, di venire incontro ai vuoti oggettivi degli organici del Servizio sanitario che naturalmente col *turnover* andranno a aumentare; cercato di non disperdere questo patrimonio, questo capitale umano importante. Devo dire la verità: in questa formulazione, per problemi tecnici, non siamo riusciti a comprendere tutte le categorie, ma lo stesso Governo ha accolto

necessità di includere tutte le realtà che hanno fattivamente partecipato all'emergenza pandemica. Pertanto, noi siamo comunque impegnati a completare questo processo virtuoso.

pandemica, ma che cerca di continuare a costruire una sinergia positiva anche col sistema del privato accreditato, che noi non vediamo come un elemento da demonizzare, ma da integrare in un'offerta che deve essere pubblica e universale.

di una norma importante, che stabilisce un primo contributo di 10 milioni l'anno dal 2022 al 2027 a favore delle Regioni per implementare questo Piano oncologico nazionale. Il ministro Schillaci in quest'Aula ha ampiamente spiegato come la prevenzione e la diagnosi precoce siano tra gli indirizzi fondamentali della sua azione di Governo; questo emendamento va in tal senso. Come vedete, si tratta di un'azione concreta, puntuale, pezzo a pezzo, che non si ferma. si ferma. Abbiamo approvato diverse norme per la proroga degli incarichi provvisori del personale sanitario e sociosanitario assunto durante l'emergenza pandemica, con la possibilità di utilizzo degli specializzanti, la possibilità di mantenere in servizio, per venire incontro alle mancanze del servizio della medicina generale di base, i medici fino a settantadue anni, soprattutto i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale, che sono stati anche decimati dal decimati dal Covid. Tanti medici sono morti perché erano la prima frontiera, erano il *front office* di un'emergenza che non si riusciva ad affrontare. È quindi logico che noi non vogliamo disperdere chi è rimasto sul campo, ma nel frattempo dobbiamo lavorare e uno degli obiettivi del Ministro della salute è quello di aumentare l'offerta dei professionisti che possono dedicarsi alla bellissima e autorevole professione sanitaria. Nel decreto-legge milleproroghe in esame abbiamo inserito diverse norme a favore degli enti locali. Ne richiamo soltanto due:

condizioni assolutamente disastrose. Il provvedimento consente di recuperare quelle risorse necessarie per mettere *in bonis* la struttura amministrativa dei Comuni che soffrono queste emergenze. Sempre in questa differimento delle adozioni dei piani di riequilibrio per i Comuni che, soprattutto a causa dell'emergenza pandemica e del caro energia (altro elemento devastante in questo momento), vivono un'emergenza finanziaria continua e costante. Concludo con un emendamento che sta molto a cuore anche a noi siciliani, a prima del senatore Pogliese, che continua a prorogare (e che sarà implementato in futuri provvedimenti) le misure a sostegno dei trasporti aerei tra la Sicilia e il resto d'Italia, perché purtroppo

non è, come detto dalla senatrice Lorenzin, un oggetto misterioso; piuttosto a me sembra una consuetudine che si ripresenta ogni anno per prorogare determinate scadenze e per introdurre disposizioni che evitano gravi problemi ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni. Una normativa di buonsenso, dunque, che abbraccia istanze promananti da tutte le forze politiche. L'esame delle Commissioni affari affari costituzionali e bilancio ne ha poi ulteriormente ampliato il contenuto, aggiungendo ulteriori previsioni, grazie a uno spirito di leale collaborazione tra maggioranza e minoranza, nonché alla sapiente guida dei presidenti Balboni e Calandrini, che ringrazio per il loro lavoro, e alla disponibilità del Governo, che ha sempre dialogato con tutti i componenti delle Commissioni per arrivare all'approvazione di ulteriori emendamenti. Nel corso dell'esame sono stati approvati 20 emendamenti a prima firma dei senatori di Forza Italia;

perché, più che nel passato, coinvolge determinati settori, quali il pubblico impiego e la sanità, spesso insieme, per garantire adeguate risorse umane a quello che è uno dei più importanti valori costituzionali, la salute dei cittadini. Sotto questo profilo, mi sia consentito congratularmi con il Governo e con le forze politiche che lo sostengono per l'evidente successo delle ultime consultazioni elettorali, che deriva evidentemente, non soltanto dai candidati proposti, ma anche da un diffuso gradimento delle azioni e degli sforzi del Governo e delle forze che lo sostengono in un contesto storico che appare agli italiani particolarmente difficile e problematico. Mi limito in questa sede a evidenziare le norme stimolate dal mio Gruppo politico e tra queste alcune fortemente caldeggiate anche dal sottoscritto, che vanno ad arricchire un impianto complessivo delineato dal Governo già di suo apprezzabile e meritevole del voto favorevole. Tornando al milleproroghe, tra le norme riconducibili all'iniziativa di Forza Italia mi limito a ricordare quelle che più incidono sui temi della sanità, del personale pubblico, della cultura, dell'energia, dell'ambiente e delle attività produttive.

per utilizzare risorse umane che sono già state formate e che hanno lavorato all'interno di questi uffici fino al 31 dicembre dello scorso anno e che hanno esperienza specifica nel settore. Come Forza Italia siamo sempre al fianco di chi lavora con impegno per tutelare e valorizzare il nostro patrimonio culturale e paesaggistico che non ha eguali al mondo. Ci aspettiamo ora che anche la fase di reclutamento prenda in considerazione queste persone, che sono formate e che erano all'interno degli uffici fino al 31 dicembre dello scorso anno. Si è prevista inoltre la possibilità per tutti gli ordini professionali - anche questo è un emendamento

Quest'anno quindi anche chi aspira ad accedere alla professione di agrotecnico, geometra o perito potrà continuare a svolgere gli esami abilitanti con le modalità semplificate che sono state adottate durante la pandemia. poi l'altro emendamento a mia firma, che propone la proroga di un ulteriore anno della durata dell'abilitazione scientifica nazionale, in modo da garantire a chi è già in possesso di quella abilitazione scientifica nella prima fascia di usufruire di finanziamenti di cui godranno le università. il differimento di altri quattro mesi della delega legislativa per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili: si capisce che oggi questi interventi di ammodernamento sono sempre più urgenti e incidono

al fine di mantenere i livelli di economicità delle attività imprenditoriali che oggi si ritrovano ad avere rincari e per fare in modo che ci sia un maggiore afflusso di clientela, perché ormai tutti preferiscono vivere all'esterno nelle città. Altri temi riguardano la sanità, la riapertura dei termini per l'iscrizione nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale, la proroga della stabilizzazione del personale sanitario, i medici di medicina generale e pediatria che saranno in servizio fino al settantaduesimo anno di età. Su queste specifiche previsioni in tema sanitario mi sia consentito di menzionare in particolare la sensibilità della nostra Capogruppo, senatrice Ronzulli, che si è spesa e ha seguito da vicino, durante queste giornate frenetiche di esame del mille proroghe, un tema delicato per il quale la sua particolare esperienza

sostiene convintamente il decreto milleproroghe e la sua conversione in legge, compresi gli arricchimenti normativi che sono intervenuti negli ultimi giorni, nella convinzione che tali previsioni consentano di affrontare le situazioni di crisi più preoccupanti.

era certamente quello delle riforme delle concessioni balneari, per dare risposte a un comparto fondamentale per il sistema turistico del nostro Paese, che da troppi anni sta vivendo una grave fase angosciante di incertezza sul suo futuro. Invece di proseguire il percorso che avevamo tracciato del riordino del demanio marittimo contenuto nel disegno di legge sulla concorrenza del Governo Draghi, che istituiva al suo interno le evidenze pubbliche per riassegnare le spiagge entro il 2024, questo Governo cosa fa? Governo cosa fa? Preoccupato di fingere di onorare promesse elettorali che non potrà mantenere, continua a non voler affrontare il tema e decide, in questo provvedimento milleproroghe, di ricominciare da capo di ricominciare da capo su un tema che era già stato affrontato, inserendo una nuova proroga - o miniproroga, come state dicendo - istituendo un nuovo tavolo con le associazioni di categoria e gli attuali concessionari. Mi rivolgo al Governo: vi rendete conto di che cosa stiamo facendo? Vi rendete conto che per l'ennesima volta stiamo portando questo settore sull'orlo del baratro, che stiamo portando il Paese ad un passo da un'infrazione europea con sanzioni salatissime

Abbiamo sempre detto che questa direttiva Bolkestein, votata da voi, quando il MoVimento 5 Stelle ancora non c'era, poteva e doveva essere trasformata in un'opportunità straordinaria, per rendere ancora più forte e competitiva la nostra offerta turistica, per portare nuovi investimenti, più sostenibilità, più servizi, più occupazione e soprattutto per avere più diritti per i cittadini, su un ma che da troppi anni viene gestito con metodo feudale e solo dalle persone che gestiscono queste aree. Per questo chiediamo immediatamente lo *stop* alle proroghe e ai privilegi e diciamo basta anche a quei concessionari che pagano 17.000 euro di canone demaniale, a fronte di fatturati da oltre 4 milioni di euro. Ce ne sono molti, famosi, nel Paese, che stanno portando avanti questo percorso. Lo dico ai cittadini fuori da quest'Aula, perché forse l'Assemblea non è attenta a quello che sta succedendo: abbiamo l'opportunità straordinaria e imperdibile di disegnare il futuro del nostro turismo balneare, ma la maggioranza di destra ritiene che invece la nostra società debba guardare con nostalgia al medioevo. Sì, parlo di Medioevo, quando vigeva la legge di quelli che erano più forti e più ricchi, che avevano più opportunità e che magari erano più furbi e senza scrupoli. Onorevoli colleghi, ancora una volta siete qui per dimostrarci che per voi governare significa piegare l'interesse della collettività all'interesse di pochi, piegare il bene comune a quello di pochi e potenti privilegiati. Noi non siamo così.

l'ennesimo tavolo sulla riforma del demanio. Signor Presidente, sa chi hanno deciso di far partecipare a questo tavolo e dunque chi decide il futuro del bene e della risorsa più preziosa per tutti i cittadini e i balneari? Non i rappresentanti dei cittadini, non i Comuni che conoscono bene le esigenze del territorio, non le associazioni ambientalistiche che tutelano gli ambienti naturali delle nostre spiagge. No,

In merito all'atteggiamento irresponsabile e inaccettabile, su questo tema, dei concessionari balneari, abbiamo presentato un emendamento soppressivo, che vuole cancellare questo vostro nuovo tentativo di perdere tempo per non decidere nulla e magari fare l'ennesima giravolta del Governo, lasciando il comparto fatto di tanti imprenditori seri, che stanno lavorando da tanti anni in maniera corretta, nella totale incertezza. Non si può perdere altro altro tempo: il Governo deve intervenire immediatamente, varare i decreti attuativi, togliere la testa da sotto la sabbia e affrontare le responsabilità nell'interesse del Paese e di tutti i cittadini.

attaccamento al lavoro, spirito di sacrificio, amore per la famiglia, per la comunità e per la propria terra: questi sono i contadini. Valori e dignità: non un fallito, ma un custode della biodiversità dei nostri territori. Fallito non è chi si laurea e decide di fare il contadino. Fallito è chi invece ridicolizza e umilia un'intera categoria e ciò è stato fatto davanti a milioni di telespettatori che pagano il canone, in prima serata, dal palco del Festival di Sanremo. Di comici che non fanno ridere il Paese ne ha avuti davvero abbastanza: va bene così. Cibo e filiera agroalimentare non arrivano dal nulla, ma dalla fatica quotidiana di oltre 740.000 imprenditori agricoli, che possiamo definire contadini. una filiera che non si è mai fermata durante la pandemia, che genera quei famosi 530 miliardi di PIL di cui tutti parlano. Nessuno ha chiesto scusa. Vi prego, facciamolo oggi da quest'Aula. Viva i laureati che scelgono di fare i contadini! Viva i contadini! *(Applausi)*. Il decreto proroga termini contiene una serie di disposizioni importanti che, grazie all'azione decisa di questo Governo, rispondono alle esigenze di enti, associazioni e categorie di aziende. Per quanto mi riguarda, ritengo incomprensibili le critiche che ho ascoltato prima al provvedimento, che ha come unico fine quello di agevolare il lavoro e l'economia. Per una certa parte politica sembra quasi che chi si sporca le mani facendo impresa, garantendo lavoro e contribuendo alla sopravvivenza e alla vita del Paese debba vergognarsi: un concetto che purtroppo qualcuno raccoglie, creando allarmismo ingiustificato e contrapposizione. Con queste misure, invece, il Governo dà un segnale di attenzione al Paese che sta investendo, seppure in un contesto internazionale difficilissimo. Passando al contenuto del decreto-legge, tante misure riguardano il comparto agricolo, che sta affrontando moltissime difficoltà. Ricordo lo slittamento dal 31 marzo al 30 giugno del termine di utilizzo del credito d'imposta riconosciuto alle imprese agricole e della pesca a parziale compensazione della spesa per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre del 2022. Inoltre, è stata estesa al triennio 2023-2025 la possibilità di incrementare del 20 per cento la quota di ammortamento deducibile ai fini Irpef a fronte di spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. È stata estesa al 2023 - questa è una misura che non è passata in legge di bilancio - anche l'aliquota di accisa ridotta per i birrifici artigianali.

l'accisa da 2,99 a 2,97 euro per ettolitro e per grado Plato. L'impatto è per i birrifici piccoli, con una produzione fino a 60.000 ettolitri, ma questa misura va anche ad aiutare i grandi birrifici che hanno un ruolo centrale nel mercato birrario nazionale, poiché sono un vero polo di sviluppo. La misura garantirà maggiore competitività alla birra prodotta in Italia, che subisce comunque una tassazione - ricordiamocelo sempre - più elevata che in Paesi come Spagna e Germania. Le accise sono tasse odiose che gravano su aziende e consumatori e colpiscono le fasce di consumatori più deboli. Sono soddisfatto che abbiamo promosso come Gruppo

sono stati poi altri interventi molto importanti. Da parte mia vorrei ribadire ancora una volta che il Governo sta rispondendo alle esigenze degli italiani con concretezza, anche con queste misure finalizzate a sostenere la ripresa della nostra economia, il cui fulcro sarà il percorso verso l'autonomia delle Regioni. L'autonomia è da sempre nel cuore della Lega, che fin dagli albori ha lottato per far comprendere l'importanza di una riforma che oggi, grazie in primo luogo all'impegno del ministro Calderoli e del vice *premier* Matteo Salvini, è diventata realtà e consentirà di far ripartire e modernizzare l'Italia, nel segno dell'efficienza, dello sviluppo e della responsabilità, a cominciare dai territori più deboli e marginali del nostro Paese. Mi permetto di chiudere con una citazione di Eisenhower: «L'agricoltura sembra tremendamente facile quando il tuo aratro è una matita e sei lontano migliaia di chilometri dal campo di grano». Questo concetto lo voglio ribadire in quest'Aula, perché vale non solo per il lavoro nei campi, ma per tutte le categorie di lavoratori. Rispettiamo sempre chi lavora; solo così non lasceremo indietro nessuno e faremo ripartire il nostro Paese.

grazie a tutto di avere così conquistato un altro pezzo di consenso; ma ho sentito usare le parole «popolare» e «rappresentanza» senza la sobrietà necessaria quando queste elezioni hanno determinato un crollo di 30 punti nella partecipazione. Non so in altre Regioni, ma penso alla mia, la Lombardia: sapere che in quella Regione dal 70 per cento delle ultime elezioni si è passati a meno del 40 per cento credo che sia un elemento che deve far riflettere tutti, perché forse questo grande entusiasmo rispetto a come si governa non è così diffuso. Lo dico come riflessione che riguarda tutti in quest'Aula, perché noi saremmo il Parlamento, che sarebbe il fondamento della Repubblica. Meno partecipazione al voto c'è, meno questo Parlamento è forte delle sue decisioni e delle sue scelte. Vorrei dedicare questo intervento non a rivendicare gli emendamenti approvati, come molti colleghi di tutti i Gruppi hanno fatto precedentemente, ma per fare alcune domande - tramite lei, Presidente al Governo e ai relatori sulle cose che un po' zoppicano invece in questo provvedimento di proroga termini, cioè su quelle cose che sono state fatte per un pezzetto, determinando condizioni di incertezza per altri lavoratori. Penso per esempio a tutti quei precari della pubblica amministrazione che godevano di un provvedimento di legge che si proroga dal 2017 e che permetteva i percorsi di stabilizzazione, quali si trovano invece di fronte al fatto che quel provvedimento non c'è più e che quindi la loro condizione di precarietà potrebbe diventare una condizione di disoccupazione. Abbiamo passato mesi a sentirci dire che era essenziale l'occupabilità e che anche l'occupabilità era di per sé una ragione per tagliare misure di sostegno, in particolare alla povertà. Ecco, vorrei che non aggiungessimo all'esercito di coloro che sono occupabili, ma che non trovano un lavoro, anche il venir meno delle certezze di coloro che invece un lavoro ce l'avrebbero e vorrebbero mantenerne le tutele. Vale, in generale, per molti dei lavoratori pubblici. Ma vorrei anche rivolgere l'attenzione al fatto che stabilizzare o meno il personale del Ministero dell'interno che si occupa delle procedure di protezione internazionale non è solo una scelta di tutela di quei lavoratori, perché non avere prorogato la protezione per gli ucraini e per i profughi ucraini nel nostro Paese si somma al fatto che le procedure ovviamente si allungano e non si danno delle risposte. Oppure vorrei dirlo rispetto ai lavoratori dell'AFAM, l'insieme delle scuole che si occupano della musica e dell'insegnamento della musica. *(Applausi)*. Vorrei ricordare che i lavoratori precari in quel settore sono quasi un quarto, non certo quindi una piccola minoranza. Eppure sono stati utilizzati degli emendamenti che puntavano appunto a prorogare la loro possibilità di stabilizzarsi e di diventare lavoratori stabili, per introdurre invece una strana norma, che ricondurrebbe i concorsi nella singola scuola e non più nel settore nel suo complesso, con uno schema che abbiamo già visto. L'abbiamo visto sull'Aifa e anche su altre cose. Guardate, non è segno di un Governo che ha un buon programma e che è pronto a governare aver bisogno del trucco di inserire piccoli emendamenti in altri provvedimenti per impedire gli effettivi processi riformatori. Lo hanno già detto i miei colleghi e lo riprendo: davvero non capisco lo chiedo nuovamente al Governo - perché la protezione per i lavoratori fragili debba essere una protezione parziale: parziale dal punto di vista che rispetto ai figli c'è nel settore privato, ma non c'è nel settore pubblico, parziale perché in realtà a coloro che non possono fare il lavoro a distanza (il lavoro agile) non riconosciamo quel trattamento ospedaliero che durante il Covid era stato pensato esattamente per proteggerli dal licenziamento. Voi sapete che tutte le normative di malattia sono regolate da un certo numero di giornate, superate le quali si va al superamento del comporto e al licenziamento. Guardate che non costa, perché, che sia trattamento ospedaliero o che sia malattia, comunque vi è un costo per le imprese e per le amministrazioni; ma in un caso salvaguardiamo la loro possibilità di continuare a lavorare, nell'altro li mettiamo a rischio. Questi sono alcuni emendamenti che avrebbero come caratteristica - qualora il Governo ci ripensasse e fosse disponibile ad accoglierli - quella di ricostruire l'insieme delle tutele che permettano a categorie di lavoratori, che sono deboli perché precari o perché fragili,

Non capiamo perché la Ministra ci ha annunciato - prima ancora che si discutesse la legge di bilancio e prima ancora che si discutesse del proroga termini - che avrebbe fatto un provvedimento e modificato la norma iniziale, perché era effettivamente e sostanzialmente discriminatoria. Quella risposta non l'abbiamo vista in legge di bilancio né la vediamo oggi nel proroga termini. La Ministra ha poi detto che lo avrebbe fatto nell'incontro con le organizzazioni sindacali, perché si sta discutendo con loro: avrebbe

ce l'abbiamo con lavoratrici che hanno già carriere contributive difficili, che raggiungono difficilmente trentacinque anni di contributi e, quando li hanno raggiunti e abbiamo comunque detto loro che la pensione sarà più povera perché sarà tutta contributiva, non vogliamo neanche dar loro il diritto di andare in pensione? Ci sono delle cattiverie, che alla fine si determinano nei confronti delle persone, che sono davvero incomprensibili. Colleghi, vorrei tranquillizzarvi: sono domande che vengono da persone che hanno dei bisogni e non una bandierina in mano hanno bisogno di avere una risposta alla loro condizione e hanno bisogno di sentirsi considerate. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che ci accingiamo a votare oggi è un importante provvedimento che contiene moltissime misure utili al sostegno del nostro sistema Paese. Tutte le misure inserite nel provvedimento di proroga termini vogliono fornire un reale supporto al nostro sistema produttivo. Per questo, il testo base del decreto-legge, così come le proposte emendative ad esso apportate, declinano un forte sostegno ai comparti italiani più significativi. Il settore agricolo, per esempio, da sempre fiore all'occhiello per le nostre eccellenze invidiate in tutto il mondo, non è secondo a nessuno né per qualità né per numeri. Nell'ultimo decennio il settore agricolo ha registrato una crescita del 10 per cento di valore aggiunto; infatti, col suo indotto alimentare contribuisce alla crescita dell'economia italiana e alla visibilità del *made in Italy* in tutto il mondo. Per questo abbiamo elaborato delle proposte per salvaguardare e preservare il settore agricolo nella sua diversità e specificità, andando a porre rimedio alle maggiori criticità e storture del sistema agricolo-economico, dovute allo stato di crisi attuale, raccogliendo rilevazioni e accogliendo proposte demandate da troppo tempo e mai - dico mai - realizzate. Rispetto alle misure inserite per il comparto agricolo, infatti, organizzazioni e associazioni di settore hanno espresso grande soddisfazione rispetto agli emendamenti del decreto-legge milleproroghe, e noi ne siamo fieri. ad esempio, all'emendamento che sostiene i produttori di birra, inserito per venire incontro a una filiera che - secondo Assobirra - conta 850 tra grandi, medie e piccole aziende, per un totale di nove miliardi di valore complessivo generato. Le stime indicano 118.000 dipendenti tra diretti e indotto e oltre 250 milioni di investimenti negli ultimi quattro anni. Ed è per loro che abbiamo voluto inserire una misura atta a ridurre il peso del fisco, limitando così il *deficit* prodotto dall'aumento delle materie prime. È quindi confermato per il 2023 il taglio delle accise sui birrifici, senza il quale per i piccoli birrifici la riduzione si sarebbe ridotta se non azzerata rispetto al 2022. Aggiungo che questa misura è stata fortemente voluta proprio per salvaguardare quel comparto storico fatto di tradizione e cultura. Anche le aziende agricole colpite da siccità, calamità e rincari energetici sono state oggetto di grande attenzione. Ci sono stati riscontri positivi anche per l'inserimento della proposta emendativa sulla possibilità

ovvero una tecnica di miglioramento genetico moderna *(Applausi)* che permette di ottenere piante resistenti ai patogeni e soprattutto resilienti ai cambiamenti climatici. Come sappiamo, negli ultimi anni le temperature medie in Italia sono aumentate; abbiamo avuto inverni miti ed estati torride; le precipitazioni hanno mutato la loro regolarità e spesso abbiamo assistito a fenomeni intensi come le bombe d'acqua. Queste nuove condizioni ambientali pongono sotto stress le attuali varietà coltivate, selezionate nel corso dei decenni per adattarsi a un ambiente che oggi non esiste più. lavorare sempre più per la programmazione e non per le emergenze. Basta emergenze. La xylella è un batterio, un patogeno invasivo che negli ultimi anni ha causato la morte e l'abbattimento di milioni di esemplari di ulivo, soprattutto in Salento, con ingenti perdite a danno degli agricoltori e di tutto l'indotto collegato. Parallelamente alla ricerca di una soluzione per il batterio, abbiamo voluto fornire un forte sostegno ad agricoltori e coltivatori colpiti dalla xylella. Spesso, infatti, si trovano a possedere piccoli appezzamenti di terreno, ma il costo per il passaggio risulta sproposito rispetto alle dimensioni. Per questo, infatti, l'emendamento proposto da Fratelli d'Italia mira a esentare il trasferimento dei terreni colpiti dal batterio della xylella da imposte catastali e ipotecarie. Questa, quindi, è una misura di supporto per facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati. Viene prorogata anche per tutto il 2023 la procedura prevista per l'emergenza Covid-19, che consente alle amministrazioni competenti di anticipare l'80 per cento dei contributi in favore delle imprese agricole, rinviando al saldo l'esecuzione degli adempimenti di verifica. Questo concede una grossa boccata d'ossigeno a tutte quelle attività in crisi che hanno necessità di liquidità e non possono soffocare a causa di una burocrazia troppo pesante e pressante. Siamo chiamati a rendere la vita più facile ai cittadini. Siamo chiamati a recepire il loro istanze e tradurle in maniera efficace per permettere loro grazie a tutto Questo è però un primo tassello, un segnale che stiamo dando a chi da tempo domanda ossigeno, supporto e sostegno, chiedendo solo di poter svolgere la propria attività all'interno del nostro sistema produttivo. un sistema che ce la sta mettendo tutta per sopravvivere. Quella climatica è da sempre etichettata come emergenza, ma emergenza non è più. Abbiamo sempre pensato che l'agricoltore abbia un basso livello culturale; invece, ogni volta che ho incontrato nella mia vita un agricoltore, ne sono uscita sempre più ricca. Mi stupiscono, conoscono l'ambiente, il territorio e le modalità di produzione. È importante sostenere l'agricoltura perché gli agricoltori saranno per noi i depositari di un patrimonio culturale.

Non c'è dubbio che il centrosinistra abbia perso le elezioni in Lombardia e nel Lazio. Ma il fatto che il 60 per cento delle persone non vada a votare desta una preoccupazione che dovrebbe interessare tutti. E forse dovremmo domandarci perché

In Commissione la maggioranza si è rifiutata di trovare 800.000 euro, e cioè meno di un milione di euro, per coprire la cassa integrazione dei lavoratori di Termini Imerese,

ma non è possibile che da un settore che produce circa 9 miliardi di reddito lo Stato abbia un incasso di 100 milioni di euro. Non è possibile: vuol dire che bisogna

di affrontare le questioni che sono sul piatto e che richiedono un intervento importante e non di aggravare la situazione esistente. È uno strumento che consente a chi governa di

Non si può che definire così l'intervento sulle concessioni balneari, uno strumento che è stato utilizzato in modo miope: prorogare *sic et simpliciter* di un anno la scadenza delle concessioni balneari significa semplicemente che tutto il comparto dei balneari resterà fermo al giorno in cui è stato già stabilito che si sarebbero dovute fare le gare, al 31 dicembre 2023, per risolvere una situazione, uno stato di fatto che ha imbrigliato il sistema; non si consente neanche ai titolari delle concessioni

senza la quale l'Italia non sarebbe riuscita a ottenere quel risultato della vaccinazione di massa che siamo riusciti a raggiungere e con la quale abbiamo superato la più grande emergenza sanitaria dal dopoguerra in avanti.

lo studente - in questo caso è stato il collega relatore - parla di tutte le cose che gli piacciono, che gli interessano e che padroneggia, tacendo ovviamente quelle sulle quali non è ferrato o che gli restano più difficili, i temi temi urticanti. Mi dispiace dunque che in questo caso il relatore abbia del tutto omesso di fare riferimento alle misure che il Governo ha inteso introdurre

sul risanamento della città di Messina. Ebbene, questa legge prevede due cose importantissime: innanzitutto, istituisce la figura del commissario straordinario governativo, individuato nella persona del prefetto di Messina, con il compito di provvedere al risanamento tramite demolizione, rimozione, smaltimento, risanamento, bonifica, riqualificazione urbana e ambientale delle aree in cui insistono le baraccopoli. Per fare questo al commissario governativo era stato dato il termine di un anno, prorogabile eventualmente di un ulteriore anno, quindi con scadenza al 31 dicembre 2022. Era stata data poi sempre al commissario governativo una destinazione di fondi importante, ben 100 milioni di euro. Se questa è la premessa, è l'intervento del Governo che sconcerta perché, alla scadenza del termine, nel momento in cui avrebbe dovuto semplicemente prorogare il tempo per l'intervento del commissario governativo affinché completasse l'opera di risanamento - stiamo parlando del ricollocamento

e non perché il Presidente della Regione non sia persona brava, professionale, intelligente e capace di fare un risanamento, ma perché ovviamente si deve occupare di tutta la Regione siciliana, mentre il risanamento richiede un impegno costante, continuo e soprattutto una presenza sul territorio che ovviamente non può garantire. Prova ne sia il fatto che ad oggi ancora non c'è stato il passaggio di consegne tra il Presidente della Regione neocommissario e il prefetto commissario uscente. Ebbene, il 1° febbraio il Governo fa un emendamento al suo stesso testo - lo presenta alle ore perché forse la sera porta consiglio - e decide semplicemente di prevedere che, affinché il commissario possa effettivamente svolgere il suo ruolo, si possa avvalere della figura del subcommissario, creando una figura in più. Ma ci serviva questa figura? No, Presidente, non ci serviva e sa perché? Il commissario, che ha già lavorato a titolo gratuito, nella persona del prefetto di Messina, ha già fatto tanto e intere baraccopoli sono già state eliminate e molta parte dei baraccati - per riferirci a loro sono stati già ricollocati, hanno avuto già modo di trovare una nuova sistemazione. Allora perché creare una figura a pagamento? Per il subcommissario, infatti, diversamente che per il commissario governativo, è previsto il pagamento di un compenso di oltre 100.000 euro. Ma non basta:

Come se questo non bastasse, il Governo fa un'ulteriore modifica, e non una proroga di termini, e prevede altresì che il commissario, che fino adesso ha lavorato per risanare, bonificare e operare riqualificazioni urbane e ambientali, utilizzi i fondi derivanti dalla partecipazione ai bandi nazionali e regionali non per riqualificare, non per costruire e realizzare veramente delle nuove aree e dei nuovi insediamenti abitativi che portino all'inclusione sociale, ma

un commissario governativo, nella persona del prefetto, ha agito in sinergia con il sindaco del Comune di Messina e con altre figure istituzionali, con Arismè, che è l'azienda speciale creata *ad hoc* per la gestione del risanamento, soggetto attuatore del commissario. invece di mantenere quella organizzazione efficiente ed efficace, si crea altro si crea un subcommissario a titolo oneroso che si avvarrà dei fondi non per riqualificare le aree urbane, ma per acquistare alloggi. alloggi. Presidente, su questo abbiamo presentato una serie di emendamenti e mi dispiace dover smentire il relatore quando ha detto che c'è stata una proficua interlocuzione con tutte le forze: gli emendamenti gli emendamenti sono stati bocciati tecnicamente, senza entrare nemmeno nel merito della discussione. Mi auguro che, dopo l'intervento di stasera, il Governo abbia modo di ripensare a quegli emendamenti e di comprendere che, se subcommissario ci deve essere,

quando già la struttura amministrativa e l'amministrazione comunale di Messina hanno dato ottima prova di sé. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, devo dire che mi sento forse la persona meno adatta a difendere il decreto milleproroghe e la discussione sulla conversione che oggi stiamo facendo. E premetto che non mi sembra questa la sede per disquisire sui risultati elettorali delle elezioni regionali. Mi sento la persona meno adatta perché considero l'istituzionalizzazione del milleproroghe una sconfitta per lo Stato di diritto, una sconfitta per la certezza del diritto; una sconfitta anche in termini educativi. È dagli anni 2000, e anche precedentemente, che ogni anno, dopo capodanno, c'è l'appuntamento ormai di prassi con il decreto milleproroghe. E la considero una sconfitta in termini educativi perché ci abitua a pensare, nel nostro Paese, che, anche se non rispettiamo i tempi, c'è sempre la possibilità di creare una proroga. Questo non aiuta a rispettare i tempi, ma soprattutto non aiuta la credibilità dell'attività legislativa che, da questi banchi, ci onoriamo di rappresentare. milleproroghe come prassi istituzionalizza dunque la fragilità del nostro sistema regolatorio. Ecco perché mi sento

mi sento di dire che abbiamo portato a casa, in un'interlocuzione positiva con le forze di maggioranza e di opposizione. Penso anche che, dal punto di vista del metodo, sia giusto riconoscere che questa è stata forse la prova di una prima interlocuzione positiva con il Parlamento. Lo dico ringraziando i Presidenti della 1a e della e il ministro Ciriani, perché forse è stata la prima volta che, in sede di conversione, abbiamo avuto lo spazio di una discussione parlamentare, che ha fatto sì che si entrasse anche nel merito dei provvedimenti. Questo lo riconosco e lo voglio riconoscere anche pubblicamente, e mi auguro che sia la prassi che vogliamo portare avanti anche per il futuro, perché - come ho sempre detto - restituisce dignità all'attività che svolgiamo in Parlamento.

mi riferisco ad alcuni emendamenti che - come sapete - sono stati presentati. Ne cito alcuni: quello sulle plusvalenze, che abbiamo visto e che poi a un certo punto è scomparso; o quelli sui diritti per le trasmissioni sportive, sui quali è evidente che c'è una diversa posizione tra alcune forze di maggioranza e tra gli stessi membri del Governo. Come ci siamo dunque comportati come Gruppo parlamentare che da sempre vuole portare avanti una battaglia di opposizione non ideologica, ma nel merito? Ci siamo dimostrati contrari a tutte quelle sanatorie che erano camuffate da proroghe *(Applausi)*, perché di sanatorie camuffate da proroghe non ne vogliamo. disponibili a discutere e a disquisire nel merito su alcune deroghe che ci sembravano necessarie e urgenti. Così è stato per l'emendamento sugli infermieri, a prima firma della senatrice Gelmini; così è stato per il tema del prezziario aggiornato per i lavori pubblici, per contrastare il caro dei materiali, senza il quale - come sapete benissimo - molte imprese costruttrici e molti lavoratori non avrebbero potuto fare i lavori, visto l'aumento dei prezzi. Così è stato con l'emendamento, a firma della collega senatrice Giusy Versace, sulla proroga dello stanziamento dei fondi di 2 milioni di euro in favore di Radio radicale. Pensate, ad esempio, che si possa andare avanti ogni anno prorogando, di 2 milioni in 2 milioni, 2 milioni, l'attività di Radio radicale? Non sarebbe molto più coraggioso dire che, quando si fa attività di trasmissione delle attività parlamentari, si svolge un servizio pubblico senza filtro, che ha bisogno di essere pagato? Abbiamo portato avanti un emendamento a firma della collega senatrice Paita in materia autostradale, chiedendo che il Parlamento tornasse a essere centrale nelle relazioni con Autostrade e non fosse ostaggio di chi ha le concessioni autostradali. È qui che si fa l'attività di confronto su un tema così delicato come le infrastrutture viarie del nostro Paese. Abbiamo portato avanti l'emendamento a firma della collega Silvia Fregolent su un tema così importante e delicato come le rinnovabili.

e ci siamo trovati a dire dei sì e dei no. Sulle proroghe camuffate da proroghe - in realtà si tratta semplicemente di prendere tempo, come sulle concessioni balneari - noi saremo sempre a favore della concorrenza. *(Applausi)*. Voi potete anche prendere tempo, ma non si può chiedere all'Europa di utilizzare i soldi del PNRR prendendo tempo, quando poi l'Europa ci chiede di fare delle riforme. Penso al tema dei precari della scuola, che è stato già citato da altri colleghi, e al tema del precariato endemico dell'Alta formazione artistica e musicale. Tutti noi abbiamo ricevuto *mailbombing*. Allora è giusto che in quest'Aula si possa dire che non si può reagire al Consiglio di Stato con una scorciatoia che non stabilizzerà il precariato endemico dell'AFAM, come volete fare con l'emendamento 6.12, sterilizzando gli Noi presenteremo un emendamento per chiedervi di togliere quella norma, perché è giusto che le persone sappiano che cosa facciamo in queste Aule *(Applausi)*. E ci prendiamo il coraggio e anche la responsabilità di dire all'esterno di quest'Aula a chi ci sta ascoltando quali sono le nostre posizioni. Presidente, forse sarò giovane e mi sarà consentito di essere un po' idealista, ma sarò contento quando, ritrovandoci all'inizio dell'anno, al prossimo capodanno - come auguro a questo Governo - o nei prossimi inizi d'anno - come auguro ai Governi che verranno dopo - non ci sarà più bisogno di votare il milleproroghe. milleproroghe. Significherà che saremo riusciti a stabilire, anzi a ristabilire, la certezza del diritto e la credibilità del legislatore,

dicembre del 2018 e alla legge di bilancio: alcuni di voi non c'erano, ma tanti se la ricordano. Il Parlamento approva la legge n. 145, dopo un periodo di trattativa tra Lega, MoVimento 5 Stelle (in quel momento erano al Governo), Forza Italia e Partito Democratico: tutti d'accordo su un provvedimento che era non una semplice proroga di quindici anni, bensì un periodo congruo per permettere a tutti di rispettare le richieste dell'Europa e per permettere ai balneari di affrontare tutte quelle novità più serenamente. Revisione del codice della navigazione, mappatura delle coste italiane, analisi sulla scarsità delle risorse, ammortamento degli investimenti, adeguamento dei canoni demaniali: tutto condiviso dai partiti che avevano lavorato alla legge n. 145 del 2018 e al decreto attuativo presentato e visto con favore dalla Commissione europea; tutto visto con favore dalle associazioni di categoria e dai tanti Comuni italiani. Come sono andate le cose lo sappiamo: il Governo Conte 2 - ce lo immaginavamo - ha disconosciuto quanto aveva approvato solo un anno prima; un anno prima il presidente Draghi andava dai balneari a ricordargli che era stato il suo Governo a fare la lasciando spazio ai detrattori, ai nuovi commissari europei, al Consiglio di Stato e ad alcuni tribunali che molto spesso si sostituiscono al legislatore. La sentenza del Consiglio di Stato, su cui poi si è basata tutta l'azione del Governo Draghi, è quanto di più sbagliato e lontano dalla realtà. I tempi dettati sono impossibili da rispettare: l'abbiamo visto immediatamente, l'abbiamo detto subito. Impossibile. La sentenza che impedisce al Parlamento di legiferare in materia è palesemente anticostituzionale. Perché è anticostituzionale? Perché la Costituzione prevede la separazione dei poteri, cari colleghi. Il potere esecutivo viene dato al Governo, il potere legislativo al Parlamento, il potere giudiziario alla magistratura. Quindi, colleghi, in quest'Aula rivendico l'indipendenza di questo Parlamento da ingerenze della magistratura. Noi rappresentiamo il popolo italiano e spetta a noi legiferare: non deve essere nessuno a dire al Parlamento cosa deve fare. Il Governo Draghi non vedeva l'ora e ha colto la palla al balzo, mettendo in difficoltà il Paese, i Comuni e il mondo del turismo balneare, usando la scusa, poi smentita, del PNRR. Io me lo ricordo: visto che c'è il PNRR, dobbiamo accelerare, per poi essere smentiti una volta approvato il provvedimento. Sappiamo tutti che il 2024 è una data impossibile da rispettare, con il rischio di mandare il Paese nel caos totale a causa di migliaia di ricorsi; e non sarà per colpa nostra. In questo decreto-legge - userò meno dei sei minuti, Presidente - abbiamo provato a mettere un'ulteriore pezza. Uno: abbiamo aiutato i Comuni a lavorare bene. Due: una mappatura seria delle coste italiane. Signori, era quanto previsto dalla legge n. 145. Presidente Draghi, era quanto previsto dalla legge n. 145. Signori della Consulta, era quanto previsto dalla Cara Europa, era quanto previsto dalla legge n. 145. *(Applausi)*. Cari colleghi di minoranza, che ai tempi avete votato e adesso criticate, era quanto previsto dalla legge n. 145. Ma avete la memoria corta: un giorno sul melo, un giorno sul pero. Colleghi di maggioranza, facciamo capire ai burocrati dell'Europa che la risorsa non è scarsa e diamo alle imprese balneari un futuro. Colleghi, dedico il mio intervento a un'amica balneare, a Patrizia, che ci ha creduto fino alla fine e fino alla fine ci ha detto: cari amici della Lega, andate avanti. E noi andiamo avanti per lei.

Signora Presidente, intervengo per farmi portavoce della grave condizione che si è registrata in Sicilia orientale a causa del ciclone mediterraneo, che, nei giorni tra il 9 e il 10 febbraio, si è abbattuto sull'isola, provocando danni ingenti, specie nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania. Si stima che solo in quarantotto ore sia caduta un settimo della pioggia che solitamente cade in un anno.

Il Sud-Est, Presidente, vive di agricoltura e proprio l'agricoltura è stata colpita fortemente in questi giorni di pioggia incessante. Investimenti per migliaia di euro sono stati travolti dal vento e dall'acqua. Il settore ortofrutticolo, già allo stremo per i rincari dell'energia e delle materie prime, rischia di subire un colpo mortale. Nel siracusano c'è la stessa identica situazione. Anche una località di grande richiamo turistico come Marzamemi è stata letteralmente sommersa dall'acqua. Nel Calatino seria la situazione di Mineo, ove anche il cimitero cittadino ha subito gravi danni, così come tutta la zona agricola dell'area a sud della Provincia di Catania. Le esondazioni dei corsi d'acqua, come a Vittoria, Lentini, Modica e Acate, hanno isolato intere zone, con problemi alle forniture idriche e di energia elettrica. Per questo motivo lo Stato ha il dovere di stare subito accanto alla Sicilia, ai cittadini, agli amministratori locali e alle imprese. Abbiamo avuto, il giorno 12, la presenza del Presidente della Regione Siciliana, insieme all'assessore all'agricoltura Luca Sammartino; abbiamo visitato insieme le zone alluvionate, cercato di dare ristoro, fatto promesse di intervento da parte dello Stato. Ringrazio pubblicamente il Presidente della Regione Siciliana e tutta la Giunta regionale per l'immediata vicinanza. Lo Stato adesso deve fare la sua parte; il Governo deve essere - e lo sarà certamente - al fianco dei siciliani, e deve farlo seguendo due direttrici: la prima è quella di intervenire con di intervenire con aiuti economici e misure di compensazione mirate; la seconda è quella di mettere in atto politiche di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico. Serve un intervento mirato; serve fare lavori come fu fatto per Genova con un commissario straordinario, per fare in modo che certe situazioni non accadano più. Troppo spesso le alluvioni distruggono i nostri territori. Sono certo che il Governo Meloni sarà al fianco dei territori del Sud, dell'ortofrutta, delle imprese e delle famiglie. *(Applausi)*.

riguarda ancora il Sud-Est della Sicilia, una zona molto fragile dal punto di vista ambientale, climatico e anche economico. nel novembre 2022 vi sono state importanti alluvioni, che hanno creato ingenti danni soprattutto al settore agricolo e a quello turistico, costringendo molti agricoltori a cambiare in corso d'opera le proprie coltivazioni. Nei giorni scorsi, per effetto dei mutamenti climatici che osserviamo e della trasformazione in eventi meteorologici estremi, ciò che avviene soprattutto in quell'area della Sicilia impatta di nuovo fortemente sulle attività economiche e sulle famiglie. Nella Provincia di Siracusa più di 70 famiglie sono state sfollate e diversi danni si sono verificati. l'impegno del Governo. Approfitto del fatto che il collega Sallemi abbia richiamato queste stesse questioni per ricordare - chiedendo l'impegno delle diverse forze politiche - un emendamento

Signor Presidente, onorevoli colleghi, senatrici e senatori, intervengo per denunciare una situazione ormai insostenibile. Faccio riferimento alla casa circondariale di Rovigo, che ebbi il piacere, con l'allora ministro Orlando, di inaugurare esattamente sette anni fa. Ieri sono stato in visita due ore e mezzo. una struttura tanto attesa e altrettanto disattesa nelle aspettative al punto che ancora manca di un direttore

sulla bocca e sulla guancia. Il dottor Alberto Burato - che mi ha autorizzato a fare il suo nome - espone questa situazione insostenibile.

chiaramente di degrado sia all'esterno, percepita appena si arriva con l'auto nei parcheggi, con immondizia dappertutto ed erba mai tagliata, sia all'interno,